Ne ha facoltà. VANO *(RC-SE)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, in questo momento, secondo le statistiche, una donna sta subendo violenza da un uomo. Il mio intervento nasce dall'esigenza di tutte le parlamentari del Gruppo della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea di tenere alta l'attenzione e la discussione sul tema della violenza sulle donne. Sia qui in Senato che alla Camera ci sentirete spesso intervenire su questa che non si può più considerare come un'emergenza, per sottrarla da tutte quelle strumentalizzazioni che l'hanno a tratti banalizzata, taciuta, o fatta scomparire.

Solo il 28 per cento dei compagni autori di violenza denunciati sono stati imputati e solo l'8 per cento condannati: il risultato è che la violenza maschile resta impunita, e non solo quella a sfondo sessuale. Dagli inizi degli anni Novanta il numero degli omicidi in Italia è diminuito di un terzo, ma il numero di omicidi in famiglia è raddoppiato: ciò vuol dire che sono diminuiti gli omicidi degli uomini sugli uomini, ma aumentati quelli degli uomini sulle donne.

che tutte finiscono con lo scomparire, col diventare altro che non violenza esercitata dagli uomini sulle donne. Queste donne però non sono altro da noi: siamo noi i milioni di bambine, ragazze, donne che ogni giorno vengono minacciate, violentate, vendute ed uccise; siamo noi le donne che si vedono negare la possibilità di reagire, quelle senza tutele; siamo noi le donne che tacciono perché non sanno parlarne o non sanno con chi farlo; noi le colpevoli di disonorare la famiglia quando denunciamo gli abusi. Vogliamo ricordare che la violenza sulle donne nasce da una cultura patriarcale e sessista e resta sempre e comunque una questione di potere. Vogliamo che non si strumentalizzi la difesa delle donne per affermare la legittimità di politiche razziste e discriminatorie. Vogliamo che le istituzioni diano soluzioni reali, credibili e coerenti per la prevenzione e la sicurezza dentro e fuori le mura domestiche. Vogliamo sempre più luoghi di accoglienza e sostegno qualificati per quante di noi decidono di raccontarsi o denunciare senza rischiare la vita. Vogliamo che gli uomini aprano una riflessione su se stessi, sul perché fanno violenza alle donne. Vogliamo che il corpo delle donne non sia più il campo elettivo di battaglie di affermazione di culture dominatrici con cui ancora, purtroppo, è difficile fare i conti. La violenza sulle donne è violenza alle donne, basta parlare di altro!

l'esame in sede referente, quindi senza mandato al relatore a riferire. In Commissione sono pervenuti molti emendamenti, presentati per la maggior parte dalla maggioranza, che hanno reso impossibile il completo esame delle proposte e la relativa votazione. Nonostante questo, il dibattito in quella sede è stato molto ampio svolto con grande correttezza e onestà intellettuale da parte di tutti, vorrei dire pacatamente, come si usa. La discussione ha evidenziato tutti i punti principali, i meriti - a nostro avviso del provvedimento ed anche le diverse posizione esistenti non solo tra maggioranza e opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza. L'opposizione, pur esprimendo giudizi critici che noi non condividiamo ha assunto un atteggiamento, nel complesso, costruttivo, di cui diamo atto. Le forze della maggioranza hanno discusso ampiamente e la sinistra della coalizione ha richiesto modifiche importanti su molti punti, punti, tenendo conto anche del dibattito intervenuto alla Camera, riguardanti l'intero equilibrio del provvedimento, il cui accoglimento avrebbe avuto ripercussioni all'interno della maggioranza e nei rapporti con il Governo e con le parti sociali, come ha rilevato in Commissione il rappresentante del Governo nella persona del sottosegretario Montagnino. Di questa situazione, quindi dell'impossibilità di superare le divergenze rilevate, si è preso atto nella fase finale del dibattito in Commissione e quindi si è pervenuti alla conclusione, che ho appena detto, di non concludere l'esame in sede referente. Insisto che il dibattito è stato privo di una conclusione formale, ma che si è svolto senza infingimenti e all'altezza dell'importanza del provvedimento.

riguarda l'origine e la legittimazione politica e sociale del provvedimento. Esso si rifà ad un accordo sociale di grande portata, che si inserisce nella tradizione della concertazione italiana e anche europea. Non è vero che la concertazione è morta in Europa; sostiene i più importanti provvedimenti sociali come esiste nella Costituzione materiale dell'Europa e come ormai è previsto nella Costituzione materiale del nostro Paese. Sottolineo questo che è un punto di prospettiva e non contingente. Nel caso specifico, questo accordo - come è noto - è stato sostenuto non solo dalla solo dalla sigla delle rappresentanze delle parti sociali, ma anche da una massiccia adesione referendaria dei lavoratori senza precedenti nella storia, che pure ha episodi simili nel nostro Paese. Sottolineo ancora, che raccoglie le istanze - proprio con questo vaglio sociale - non solo del mondo del lavoro, ma del mondo produttivo, con vari provvedimenti noti ai colleghi e che quindi non non cito. Riguardano le istanze del mondo del lavoro e della produzione non solo del settore industriale, contrariamente a quanto hanno detto alcuni alcuni colleghi dell'opposizione, perché anche il mondo dei servizi e delle piccole imprese è stato considerato con provvedimenti specifici. Il secondo punto generale che intendo evidenziare perché anche questo ha un rilievo di prospettiva - riguarda i rapporti tra Governo, parti sociali e Parlamento. Si tratta di un punto molto dibattuto, critico, nelle esperienze non solo italiane. Il Governo, come è noto, ha ritenuto di riprendere sostanzialmente i contenuti del Protocollo del 23 luglio scorso, poi negli aggiustamenti successivi - sappiamo quanto sia stato difficile l'*iter* - ha tenuto conto di richieste di modifica provenienti anche da varie forze politiche che si sono

duplice esigenza di essere fedele all'accordo sociale, senza però essere insensibile alle richieste delle forze politiche. Questi aggiustamenti non sono anomali: anomali: nella storia della concertazione italiana si sono riprodotti episodi del genere. Nel nostro caso specifico, come è noto, tali aggiustamenti sono stati particolarmente sofferti, non tanto per il merito di singoli punti, pure importanti, come i lavori usuranti ed i rapporti a termine, che toccano delicate questioni del mondo del lavoro, ma in realtà proprio per la difficoltà e la delicatezza degli equilibri politici

che l'intero equilibrio venisse sottoposto ad una verifica politica all'inizio di gennaio. Tutto ciò ha evidentemente pesato nel dibattito in Commissione,

di carattere istituzionale. Si è discusso a lungo delle prerogative del Parlamento e del rapporto - appunto - tra Governo, accordo sociale e decisione finale. In realtà, questione è molto chiara, sia nella prassi italiana che in quella di altri Paesi: è evidente che in un processo di concertazione, che richiama esigenze di governabilità, il ruolo dell'Esecutivo è essenziale, in quanto è il Governo che si assume la responsabilità di tradurre i contenuti dell'accordo in un provvedimento finale avente forza di legge, ponendo alle forze di maggioranza un vincolo che ha diversa stringenza a seconda delle

Proprio la gravità e l'importanza di questa posta in gioco ed il valore complessivo di grande rilievo del Protocollo inducono ad affrontare il dibattito con la ferma convinzione che il provvedimento in esame una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Treu, il disegno di legge n. 1903, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo del proponente, senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del nostro Regolamento.

è di fondamentale importanza perché attua il Protocollo del 23 luglio 2007, frutto di un processo democratico che ha visto circa 5 milioni di lavoratori e pensionati aderire al *referendum* indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e approvare l'accordo. Il testo che oggi esaminiamo raccoglie le necessità e le esigenze espresse da quei lavoratori che hanno visto in questa potenzialità

che spesso ostacola la realizzazione di un progetto di vita familiare e sociale. Il provvedimento tiene conto di tutti questi aspetti e, in particolare, affronta

Questo scalone produceva una evidente ingiustizia, un'ingiustizia che riguardava circa 130.000 lavoratori che il prossimo anno, dal 1° gennaio, si sarebbero trovati bloccati bloccati dall'aumento improvviso e subitaneo dell'età minima fissata in sessant'anni. Con il disegno di legge oggi al nostro esame si elimina questo scalone e si prevede una maggiore elasticità combinando insieme l'età anagrafica e gli anni di contribuzione. Credo che questo rappresenti un passaggio importante che certamente ha un costo rilevante per le casse pubbliche, non solo per il prossimo anno ma anche per gli anni futuri, ma è un modo per dare certezza e le certezze nel campo previdenziale sono un elemento essenziale.

da poter giungere al superamento delle diffuse situazioni di precarietà. La parola chiave che soggiace a questa parte dell'accordo è l'ambizione di voler tramandare ai nostri ragazzi la possibilità di dimostrare sul campo la loro competenza e di poter vedere nel loro futuro non solo incertezza e precarietà, ma anche qualche sicurezza e orizzonti meno incerti. Attraverso la delega legislativa si potenzia, infatti, il sistema d'incontro tra domanda e offerta di lavoro semplificandone le procedure si abolisce l'istituto del lavoro intermittente o a chiamata, cosiddetto *staff leasing,* spesso utilizzato come forma di lavoro senza alcuna garanzia per i giovani lavoratori. Per ciò che concerne i contratti a termine, nel caso di una successione di questa tipologia di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti, se il rapporto di lavoro avrà superato complessivamente i trentasei mesi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, tale rapporto sarà considerato lavoro a tempo indeterminato. Vengono inoltre previste risorse per lo svolgimento di attività innovative e imprenditoriali per consentire l'accesso al credito a chi ha meno di venticinque anni e per sostenere i compensi, cioè la retribuzione, durante lo svolgimento di attività lavorative intermittenti. Si stanziano 24 milioni di euro per tre anni (2008, 2009 e 2010) a sostegno dei giovani ricercatori universitari, titolari di assegni e contratti di ricerca. Si introduce la possibilità di di cumulare periodi assicurativi riferibili a differenti gestioni pensionistiche (la cosiddetta totalizzazione) e di riscattare la laurea a fini previdenziali. Si prevede altresì la possibilità di detrarre a fini fiscali dal reddito dei genitori o del soggetto di cui si è fiscalmente a carico il costo dei contributi riscattati, nel caso in cui il giovane non abbia ancora un reddito personale tassabile;

di avere invece un sistema di copertura previdenziale dignitoso e corrispondente all'insieme della loro carriera di studio e lavoro. Un'ultima osservazione: credo che questo accordo ponga le basi anche per una revisione sostanziale del *welfare*, con uno sguardo più decisamente rivolto al futuro. Vi sono due parti, nell'accordo appena accennate, che dovrebbero diventare il cardine di un*welfare* dell'opportunità e della nuova protezione sociale. Esse riguardano, da un lato, la necessità di introdurre il diritto alla formazione permanente, come costitutivo del diritto del lavoro e nuova forma di tutela del lavoro nella società della conoscenza. A questo proposito, vi è già uno schema di disegno di legge del Governo,

per le generazioni future, coloro che già lavorano o sono in cerca di un lavoro. Dall'altro lato, in questo accordo rimangono sostanzialmente in ombra le nuove forme di protezione sociale, che riguardano la politica familiare,

del Senato) il rischio che la protezione sociale sia pensata unicamente o totalmente in forme individuali, lasciando da parte il fatto essenziale che le persone vivono in nuclei familiari, potrebbe generare nuove diseguaglianze e disequità e, soprattutto, non consentire una piena e completa conciliazione tra il lavoro e la vita professionale. L'annunciata verifica di gennaio non può non porre questi due temi in cima alle priorità di un Governo che voglia realizzare un impegnativo programma di riforme, sostenendo e promuovendo, in particolare, le condizioni segnate da maggior debolezza e rimuovendo le cause dell'esclusione sociale di tanti nostri cittadini. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il cosiddetto scalone è la più pesante eredità, sul piano sociale, lasciata dalle destre al Paese e ai lavoratori. Dopo la riforma della legge elettorale, questa è la seconda provocazione fatta sulla pelle degli italiani che il Governo Berlusconi, ormai in declino, ha voluto lasciare alla maggioranza che sarebbe subentrata (ed è stata di centro-sinistra). Meriterebbe una riflessione un atteggiamento che prevede di scaricare fuori dall'arco temporale della propria competenza norme e proposte che non incontrano alcun consenso nel Paese, segno di una grave irresponsabilità politica e istituzionale. La scelta di prevedere una differenza nei diritti delle persone così profonda, La scelta di prevedere una differenza nei diritti delle persone così profonda, tre anni di lavoro in più o in meno, che maturasse nell'arco di una notte, era insostenibile e inaccettabile. Purtroppo, alla provocazione confezionata dal Governo Berlusconi il provvedimento in esame, sul terreno pensionistico, risponde in modo assolutamente insoddisfacente. Questo giudizio non inficia il rispetto che abbiamo per l'autonomia delle forze sociali che hanno sottoscritto il Protocollo, ma tale rispetto non può giustificare il *vulnus* che si è prodotto alla Camera dei deputati, cioè la limitazione della libera espressione della volontà del Parlamento, eletto senza vincolo di mandato, come recita la nostra Costituzione. Questo accordo certamente abolisce l'iniquo scalone ma, seppure con maggiore gradualità, alza pesantemente l'età pensionabile, costringendo uomini e donne, che sulla loro fatica hanno costruito la ricchezza del Paese, a prolungare l'attività lavorativa. Neppure si è scelta la via dell'innovazione, come sarebbe avvenuto differenziando l'età pensionabile a seconda del tipo di lavoro che ciascuno ha svolto nel corso della vita. La timida e povera proposta che riguarda i lavori usuranti non risponde a questa esigenza, limitandosi a cedere alle pressioni fatte dalla parte più arretrata del mondo imprenditoriale. Nei giorni scorsi abbiamo assistito ad una discussione inquinata da argomenti strumentali. Il dato che l'INPS sia tuttora gravato da costi assolutamente estranei alla materia pensionistica, come le spese di assistenza sociale, è incontrovertibile, come è incontrovertibile che il fondo dei lavoratori dipendenti oggi stia pagando le pensioni di fondi in rosso come quello dei *manager*. Una curiosa forma di solidarietà al contrario. Un ultimo caso, deciso poche settimane fa, è stata la scelta di scaricare sull'INPS e sull'INAIL il fondo degli sportivi, la SPORTASS, che aveva ormai accumulato 170 milioni di debiti. Se questo è lo stato rispetto alla materia pensionistica, ancora peggiori sono state le decisioni prese in materia di lotta alla precarietà per timidezza ed inefficacia. Nella società che cambia, alcuni vorrebbero che la precarietà diventasse un dato strutturale su cui fondare la competizione internazionale, perché è più facile per una impresa, che si occupa più di rendite che di prodotto e che non ha il coraggio dell'innovazione, riversare le proprie debolezze sul costo del lavoro e sulle condizioni di vita dei lavoratori. Questa è la posta in gioco: o una società fondata sulla conoscenza, sull'innovazione, sulla competizione alta, oppure una brutta copia delle tigri asiatiche, dove i lavoratori sono soggetti senza diritti né futuro, e la sicurezza un costo da eliminare dal bilancio con un tratto di penna. Davanti a tale alternativa, il Governo ha rinunciato a decidere, delegando alle imprese il modello di sviluppo del Paese; un'abdicazione grave. Ha abdicato non solo quando ha deciso che tre anni non sono sufficienti per avere un lavoro stabile, con un futuro davanti, ma anche quando ha rinunciato ad affrontare la condizione dei più precari tra i precari: Co.co.pro., interinali, assegnisti, borsisti. È su questo che, alla Camera dei deputati, il Governo ha scelto di zittire la propria maggioranza, ponendo la fiducia su un testo diverso da quello approvato in Commissione lavoro, che con un apprezzabile sforzo, pur senza contraddire i contenuti del Protocollo, migliorava i punti di maggiore sofferenza. Ancor di più, dopo le inadeguatezze contenute nel provvedimento che stiamo esaminando, salario e precarietà saranno i temi sui quali sarà misurato il Governo. È tempo di dimostrare di saper aggredire e risolvere i problemi sociali più drammatici del nostro Paese. *(AN)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, mi soffermerò su tre aspetti che riguardano il disegno

il metodo, ha già detto il presidente Treu che il provvedimento arriva in Aula senza relatore. Aggiungo, per informazione dei colleghi, che giunge in Aula senza l'esame

si è detto, anche negli interventi di coloro che mi hanno preceduto, che questo doveva combinare le giuste aspettative degli anziani con le giuste speranze dei giovani. Basta fare una piccola contabilità intergenerazionale per capire che gli anziani non sono certo fortemente agevolati e i giovani continuano ad essere fortemente penalizzati. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, in ogni Paese civile del mondo occidentale la contabilità intergenerazionale è uno strumento che viene messo a disposizione del Parlamento, in modo tale che i rappresentanti del popolo possano conoscere le conseguenze dei provvedimenti che vanno a votare, capendo prima come queste producano effetti non solo tra di noi, cioè nella generazione al comando del Paese - normalmente quella che sta oltre i cinquant'anni - ma soprattutto nelle generazioni successive. Ci sono fior di studi su questo aspetto: in Italia tale metodo è entrato più recentemente, ma ho la sensazione che possa essere a perfetta conoscenza di diversi rappresentanti del Governo,

soprattutto in termini di *welfare* e mercato del lavoro, dell'impatto tra le diverse generazioni. Ma ciò che conta, nel merito del provvedimento, è che in realtà per spalmare lo scalone e ridurlo in scalini si è caricata la nuova generazione di circa 10 miliardi di euro in più di debito sulle spalle. Questa è la sostanza del provvedimento, cioè una redistribuzione socialmente iniqua che dà un piccolo vantaggio di ritardo nel pensionamento della nostra generazione e carica questo costo sulla generazione dei giovani, cioè di tutti coloro che sono entrati nel mercato del lavoro dopo il 1995, che sono già a regime di ripartizione contributiva, che sanno già che avranno una pensione pari al 35 per cento del loro reddito. Quindi carichiamo un debito su chi avrà una pensione pari al 35 per cento della media dei loro stipendi futuri per dare una piccola agevolazione di ritardato pensionamento alla generazione ancora a regime di ripartizione retributiva, quindi al livello massimo di regime pari a quarant'anni di contributi, all'80 per cento della pensione rispetto alla media delle ultime retribuzioni, la più perversa delle redistribuzioni sociali del reddito in termini intergenerazionali.

di far sì che il Parlamento, in questo caso il Senato, conoscano esattamente ciò di cui stiamo parlando. In Commissione bilancio, giusto ieri, è emerso un aspetto fondamentale del provvedimento rispetto al quale, senza un chiarimento del Governo, non so cosa i colleghi senatori voteranno, sia che si esprimano a favore, sia che si esprimano contro il provvedimento. La questione riguarda i lavori usuranti ed il trucco parallelo, che è stato in qualche modo utilizzato nel caso, che abbiamo affrontato la settimana scorsa, della stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione. Ci sono due numeri che non quadrano.

Il Governo deve dire con grande trasparenza e franchezza al Parlamento e al Senato, e possibilmente con urgenza (è soprattutto il Ministero dell'economia, che in questo caso deve fare queste valutazioni),

mansioni usuranti che il provvedimento in realtà determina supera di gran lunga le 5*.*000 unità, qualcuno immagina 20.000, allora il provvedimento è palesemente privo di copertura*.* Questo elemento*,* signor Presidente, non èemerso nella *buvette*, non è emerso nei corridoi del Senato, ma ieri in Commissione bilancio, tanto che il parere della Commissione sulla copertura

In base a tale dato la Commissione bilancio ha potuto rilasciare il proprio parere, senza comunque aver discusso gli emendamenti. Ma, giustamente e legittimamente, un membro della Commissione della maggioranza ha votato contro questo parere, perché ha sostenuto, correttamente e giustamente dal suo punto di vista, che quel numero di 5.000 non c'è

chiedo formalmente al Governo di venire in Aula, possibilmente all'inizio di questa discussione generale, altrimenti non si capisce di che cosa parlino i colleghi della maggioranza e dell'opposizione, trattandosi di un provvedimento per il quale non si sa

dopodiché, con 20 milioni di euro si possono però stabilizzare non più di 3.000 precari e tutti hanno sostenuto che i precari sono 350.000. allora, delle due l'una: o i 350.000 vinceranno i ricorsi, quindi quel provvedimento invece di costare 20 milioni di euro, costerà 5-6 miliardi sempre a carico poi delle nuove generazioni, oppure non si stabilizzeranno ed in questo caso è una clamorosa ipocrisia e bugia quella di dire che i precari della pubblica amministrazione, seppur nel tempo, verranno stabilizzati. Qui siamo di fronte esattamente allo stesso problema, signor Presidente.

nel provvedimento o comunque non è chiarito dal Governo, siamo palesemente di fronte ad una norma priva di copertura. Non lo dice soltanto il senatore Baldassarri in questo momento in Aula, ma è la sostanza di quanto è stato ieri alla Commissione bilancio da un senatore della maggioranza che ha giustamente, dal suo punto di vista, almeno in modo trasparente, sollevato l'argomento.

Signor Presidente, come già evidenziato in precedenza, il provvedimento che siamo chiamati ad esaminare recepisce il Protocollo dello scorso mese di luglio, sottoscritto tra quasi tutte le parti sociali e il Governo. Un Protocollo sul quale si sono pronunciati oltre cinque milioni di lavoratori e di lavoratrici, marcando un vasto consenso sui contenuti del documento. Si è dato luogo, in quell'occasione, a una grande prova di democrazia da parte delle organizzazioni sindacali: un avvenimento straordinario che qualifica il tasso democratico di tutto il nostro Paese. In via generale, il presente provvedimento, che raccoglie appunto i contenuti di quell'accordo, s'inserisce a pieno titolo nell'alveo di una serie di interventi che hanno distinto l'azione del Governo e della maggioranza nell'arco di questi diciotto Si è lavorato, infatti, per affermare una politica economica a sostegno della crescita e dello sviluppo del Paese, realizzando un positivo abbassamento del debito pubblico, favorendo la crescita del PIL (la più alta registrata negli ultimi sei anni), consolidando il rilancio complessivo del nostro sistema economico, dimostrato per altro dalla stessa ripresa delle esportazioni. Nel complesso, quindi, il disegno di legge in esame si caratterizza, a mio parere, per due elementi di fondamentali importanza nel contesto sopra richiamato: mette a regime il sistema pensionistico, determinando una condizione di stabilità che nei prossimi anni eviterà di dover riprendere costantemente il tema delle pensioni; e, in secondo luogo, mette in campo una serie di misure e di provvedimenti volti a rendere più stabili e meno precarie le prestazioni lavorative, in un mercato del lavoro che pure sappiamo essere ormai quasi strutturalmente caratterizzato da una necessaria flessibilità. Da questo punto di vista, vorrei ricordare che le misure contenute nel provvedimento sul versante della lotta alla precarietà e della stabilizzazione dei rapporti di lavoro si collegano strettamente ad una serie di altri interventi che nel corso di questi mesi hanno visto protagonista l'azione del Governo. Azione ha segnato un particolare impegno del Ministro competente, a partire dagli interventi per dare copertura ai diritti di malattia e maternità dei lavoratori a progetto, fino ai provvedimenti assunti con le parti sociali volti a stabilizzare circa 23.000 lavoratori di *call center*.

si può fare di più, e lo si dovrà fare, su questo delicato versante. In ogni caso, sarebbe un grave errore non considerare l'opportunità e la necessità di dare corso all'approvazione del presente disegno di legge, valutata, in particolare, la scadenza ormai vicina del 31 dicembre 2007, data che segna l'eventuale entrata a regime della cosiddetta riforma Maroni e, conseguentemente, del tanto discusso «scalone». Una riforma del sistema pensionistico promossa dal precedente Governo senza alcun confronto con i soggetti interessati, determinando, fra l'altro, una vera cesura tra generazioni di lavoratori e lavoratrici, a scapito, in particolare, di quelli più giovani. Da questo punto di vista, quindi, e per la prima volta, il provvedimento, che recepisce il Protocollo di intesa, non si occupa soltanto dei padri, ma si occupa in modo consistente anche dei figli. In particolare, si propone decisamente il superamento dello «scalone», senza però rinunciare all'esigenza strutturale di allungare l'età pensionabile, e ciò viene fatto in modo più graduale, tenendo conto delle specificità di condizione di lavoro di chi, nell'arco della propria vita lavorativa, è stato sottoposto ad una prestazione usurante sul piano fisico o su quello psichico. Si attua poi un consistente intervento volto ad aumentare le pensioni più basse, in una situazione nella quale, per altro, è posta all'ordine del giorno l'attenzione sul delicatissimo tema del necessario adeguamento dei salari e delle pensioni di fronte alla crescita del costo della vita. In via generale, la soluzione individuata tiene conto dell'esigenza di chiamare tutti i lavoratori e le lavoratrici, e non solo una parte di essi, a sostenere gli oneri connessi all'equilibrio del sistema previdenziale. Sempre su questo versante, va evidenziato ancora che il presente provvedimento prevede significative misure riguardanti la totalizzazione dei periodi contributivi, versati in qualsiasi modalità e tempo lavorativo, e il riscatto degli anni di studio universitario. Entrambe queste misure, come risulta del tutto evidente, sono volte a favore delle giovani generazioni, che guardano oggi alla propria vita lavorativa con preoccupazione ed incertezza sul futuro. Segnalo poi all'attenzione dell'Aula gli interventi volti ad avviare la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Una riforma che si propone - badate bene - in una chiave finalmente «universalistica», superando l'impostazione di natura assistenziale, per realizzare così uno strumento che sia funzionale alle nuove tipologie contrattuali, con il concorso dei servizi per l'impiego, in un contesto di forte, proprio forte collaborazione fra Stato, Regioni e parti sociali. In questo quadro, gli obbiettivi principali sono fissati con l'adozione da parte del Governo di uno strumento unico, volto al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati, nonché con la previsione di contribuzione figurativa, ai fini previdenziali, per chi beneficia dei trattamenti di disoccupazione. Ma ancora (e credo che ciò vada segnalato con forza), il presente disegno di legge si propone di consolidare tutte le misure a sostegno e a favore dell'occupazione femminile, introducendo in particolare la stabilizzazione dei contratti a tempo indeterminato per le donne. Meritano, infine, precisa attenzione gli interventi volti a consolidare il sostegno alla competitività delle imprese, come la riduzione della tassazione sul salario di produttività e le misure che integrano la riduzione del cuneo fiscale, prevista anche quest'anno nella legge finanziaria. Vi sono pertanto, a mio avviso, molte ragioni per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, che indubbiamente recepisce fondamentali richieste provenienti dal mondo del lavoro. È chiaro, però, che l'impegno del Governo e della maggioranza sul versante sociale non potrà esaurirsi con il varo delle norme che recepiscono il Protocollo del 23 luglio. In particolare, dovrà essere affrontata con decisione la questione salariale e attuati ancora con più forza e determinazione gli interventi necessari a promuovere una crescita sostanziale della produttività del nostro sistema Paese. Sul fronte salariale, va ricordato l'impegno anche di questo ramo del Parlamento: impegno che si distingue con l'avvio di un'indagine conoscitiva, da parte delle Commissioni 6a e 11a riunite, per approfondire i profili contributivi e fiscali del problema. In ogni caso, la questione concernente il livello dei salari e degli stipendi e la difesa del loro potere d'acquisto è oggi con forza, come dicevo, alla nostra attenzione. Si tratta di lavorare, pur nel rispetto dei rispettivi ruoli, chiamando a responsabilità tutte le parti sociali, a cominciare dai rappresentanti delle imprese, per dare corso rapidamente, ad esempio, al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Sul fronte relativo al fisco, ai prezzi, insomma al potere d'acquisto di stipendi e salari, risulta non più rinviabile una decisa azione da parte del Governo e della maggioranza affinché s'intraprendano celermente una serie di interventi che offrano la possibilità, alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, di affrontare con più tranquillità gli impegni del quotidiano e del futuro. Concludendo, signor Presidente, voglio far presente che su questo contesto di problemi la legge finanziaria annuncia prime importanti misure, che andranno realizzate già a partire dall'immediato futuro, con riferimento in particolare alla possibilità di dedicare eventuali maggiori entrate fiscali a favore della riduzione della tassazione sui salari. *(UDC)*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, prima di passare all'analisi della portata economica e sociale del Protocollo sul *welfare*, ritengo opportuno svolgere una premessa di ordine politico. Molte delle considerazioni che andrò a svolgere sono state già anticipate in Commissione e credo che saranno riprese nel corso del dibattito. L'esproprio delle prerogative parlamentari di quest'Aula, infatti, come del resto quelle della Camera pochi giorni addietro, è un fatto evidente ed ormai di dominio pubblico. Vale la pena, tuttavia, sottolineare lo sconcertante gioco delle parti che il centro-sinistra è riuscito a imbastire nell'approvazione di questo Protocollo sul *welfare*. Inizialmente, il Governo ha elaborato il testo di concerto solo con i sindacati e l'associazione degli industriali, lasciando fuori importanti settori del mondo economico e imprenditoriale: basti pensare all'inaccettabile disparità di trattamento tra lavoratori autonomi e dipendenti, fino a pericolose fratture tra questi due mondi. Quel testo che Quel testo che - giova ricordarlo - doveva essere intoccabile, provocò una situazione assurda: da una parte si aderiva al Protocollo con un*referendum* votato dai lavoratori appartenenti ai sindacati che avevano sottoscritto un patto con il Governo; dall'altra, insorgevano i parlamentari della sinistra radicale, quella che, pur sentendosi più vicina alle organizzazioni sindacali, decideva di manifestare contro gli accordi da loro presi con il Governo. La frattura, che sembrava insanabile, si ricompose temporaneamente solo attraverso la proposizione in Aula alla Camera del maxiemendamento, sul quale venne poi imposta e votata la fiducia. Il fatto provocò allora le dimissioni dell'onorevole Pagliarini, presidente della Commissione lavoro, in aperta polemica con il Governo, colpevole, a suo dire, di non aver voluto rispettare il ruolo istituzionale del Parlamento. Le dimissioni, ieri rientrate, vista la sua pronta rielezione, costituivano un evidente gesto simbolico, cui il Governo si è comunque mostrato sordo. si è ripetuta la stessa farsa: la Commissione lavoro non ha potuto esaminare alcun emendamento a causa dell'ostruzionismo manifestato dai senatori della sinistra, che ha di fatto reso impossibile la discussione. Ed oggi il testo arriva in Aula, senza relatore, nell'evidente imbarazzo di una maggioranza ormai lacerata, sostenuta solo da una logica di mera sopravvivenza. Il fatto sconcertante non è tanto l'ennesimo voto di fiducia che qui verrà richiesto, quanto piuttosto l'assurdo paradosso che è sotteso a questo atteggiamento. L'ostruzionismo dei lavori parlamentari, infatti, è di solito posto in essere dall'opposizione al fine di ritardarne il corso. Credo sia una novità assoluta quello posto in essere dai parlamentari di una parte della maggioranza, quella che viene chiamata democratica: questi, infatti, presentano un numero impressionante di emendamenti ad un testo che il loro Governo ha deliberato con le parti sociali; sanno che è blindato e quindi intoccabile; sanno che non ce ne sarebbe neanche il tempo, vista la scadenza della legge Maroni, che a qualsiasi prezzo intendono modificare. Ma di questo a loro non importa nulla, perché la loro azione si riduce al solo scopo di impedire che vengano discussi quegli emendamenti presentati da un'altra parte della maggioranza, quella che viene chiamata radicale. La prima non può permettersi il confronto con le proposte della seconda in materia di lavoro, pensioni e *welfare*, ma ha bisogno del suo voto per sostenere, non il Governo della maggioranza elettorale degli italiani, non il Governo di una maggioranza parlamentare, ma quello solo di una parte della maggioranza. Da un lato, vi sono parlamentari che paventano la crisi di Governo e, pur di evitarla, espropriano il Parlamento di fatto, prima ancora che di diritto, di ogni sua prerogativa costituzionale; dall'altra, parlamentari che vengono costretti a rinunciare al responsabile esercizio del proprio mandato, perché impossibilitati a discutere ed emendare un disegno di legge fondamentale per le prospettive sociali ed economiche della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, siano essi lavoratori, imprenditori, giovani in cerca di lavoro o anziani che vogliano concludere dignitosamente la propria carriera. Allora sorge spontanea la domanda: possibile che la tutela dei lavoratori, e dei cittadini italiani tutti, venga subordinata alla vostra paura di perdere le prossime elezioni? La vostra azione politica, alla fine, tolte tolte tutte le sceneggiate e le rivendicazioni, le questioni morali e quelle di principio, si risolve solo in questo: evitare la crisi di Governo e il ricorso alle urne. Nell'evidente consapevolezza del sentimento negativo che ormai avvolge la vostra coalizione, avete bloccato una Nazione. La paura vi ha paralizzato e conseguentemente ha paralizzato tutta l'attività istituzionale. Nelle Aule parlamentari, come in quelle di Commissione, non solo non si producono più leggi, ma non si discute neanche più alcun testo, riducendosi tutto in un avvilente gioco delle parti dove la sopravvivenza del Governo è l'unica trama. Arriviamo così a parlare del famigerato contenuto di questo testo, che ha il privilegio di non essere stato discusso né emendato in alcuna sua parte, né alla Camera né al Senato. Non fosse altro per l'indubbio onore della cronaca che a questi interventi riserva ormai solo il Resoconto stenografico. Se l'approvazione da parte vostra di questo disegno di legge soggiace alle vostre paure, il suo contenuto invece si appiattisce sulla vostra ormai arcaica concezione del mondo del lavoro. Le promesse fatte in campagna elettorale andavano mantenute e l'abolizione della riforma Maroni e della legge Biagi rappresentavano da allora quell'obbiettivo fondamentale da cui la vostra stessa sopravvivenza politica sembra non poter prescindere. E questo a discapito di ogni realistica quanto lucida analisi della realtà economica e sociale. Innanzi tutto, vale la pena ricordare le ingenti spese che investono il bilancio previdenziale a causa della revisione dello «scalone». Per consentire a poche decine di migliaia di lavoratori, peraltro non stressati né usurati, di anticipare il pensionamento, si sono addossati con l'aumento delle aliquote contributive nuovi oneri alle giovani generazioni, a tutto discapito di tanta retorica sull'equità tra le generazioni. Vi siete infilati nel vicolo cieco dell'abolizione dello «scalone», lo avete sostituito con gli «scalini», ma non vi siete mai soffermati a chiedere quali fossero i costi sociali di questa abolizione. Continuate poi a ripetere la vostra assoluta contrarietà nei confronti della legge Biagi, a discapito di tutte le analisi economiche che ne evidenziano i benefìci, dando la disoccupazione ai minimi storici. E, pezzo dopo pezzo, la state svuotando. La vostra miopia vi impedisce di fare un'analisi lucida della situazione. Spesso vi siete anche contraddetti: avete affermato che lo *staff leasing* e il lavoro a chiamata fossero una tipologia di lavoro precarizzante; poi avete cercato di reintrodurre almeno il *job on call*, perché la sua reintroduzione sarebbe servita ad impedire a tanti lavoratori di ricadere nel sommerso. Ma allora delle due l'una: o sono istituti precarizzanti o sono istituti posti a tutela dei lavoratori. La vostra onestà intellettuale si perde nel gioco delle parti che siete costretti a sostenere. Invece, si sarebbe potuto analizzare insieme la reale situazione prodotta dall'applicazione della legge Biagi: avremmo potuto integrarla con ammortizzatori sociali più validi e più attivi; così facendo, avremmo insieme garantito al Paese le condizioni di un mercato del lavoro moderno e competitivo, flessibile ma garantito. Invece, da soli andate avanti seguendo a tutti costi un programma elettorale che l'onorevole Giordano ha definito, nel suo intervento alla Camera dei deputati, «pura archeologia industriale». Non possiamo inoltre accettare che con un voto di fiducia venga stabilita la disparità di trattamento fra lavoratori autonomi e dipendenti per quanto riguarda tutti i punti salienti del vostro Protocollo, l'età di accesso alle pensioni di anzianità e per le finestre di pensionamento, ma soprattutto per l'assurda esclusione dai lavori usuranti. Né possiamo accettare che venga rimandata a criteri vaghi, discrezionali ed ambigui la definizione della categoria dei lavoratori usuranti. In chiusura, mi permetto di esternare un ultimo commento sulla razionalizzazione degli enti previdenziali. Abbiamo già più volte espresso il nostro parere contrario non solo sulla sostanza del provvedimento, ma anche sulla possibilità che possa essere fonte di rilevanti risparmi; risparmi che nel testo vengono dati per certi, pure in mancanza della presentazione di un piano industriale. Le coperture previste (3,5 miliardi di euro) già oggi appaiono precarie; se si deve poi prevedere una clausola di salvaguardia in base alla quale, se non si registreranno i risparmi ipotizzati, scatterà a partire dal 2011 un ulteriore aumento contributivo generalizzato dello 0,09 Ormai è chiaro che vi sono troppi elementi, nel vostro Protocollo ed in questo testo oggi in esame, che danno la misura di una concezione centralista e assolutamente sbagliata del mondo del lavoro.

Signor Presidente, anch'io vorrei sottolineare che il disegno di legge all'esame dà attuazione all'accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, un provvedimento che riguarda una serie di materie che vanno dalla previdenza al mercato del lavoro, agli ammortizzatori sociali, alla competitività, all'inclusione sociale, in un'ottica di crescita e di equità. Nei che scaturisce dalla concertazione adottata dal Governo come asse portante delle politiche sociali e del lavoro. Si tratta il disegno di legge in esame prevede interventi volti a realizzare migliori condizioni previdenziali e lavorative. I risultati di maggiore spicco riguardano, in particolare, la modulazione graduale dell'età pensionabile rispetto al cosiddetto scalone, una modulazione che determina una condizione di maggiore equità, tiene conto della condizione di lavoro di coloro che svolgono attività usuranti ed evita che problemi di equilibrio della spesa previdenziale vengano posti a carico esclusivamente dei lavoratori dell'industria, addetti, in molti casi, a mansioni pesanti e nocive. La soluzione individuata con il disegno di legge all'esame tiene infatti conto dell'esigenza di chiamare tutti i lavoratori, e non solo una parte di essi, a sostenere gli oneri connessi all'equilibrio del sistema previdenziale. Sempre sul versante previdenziale, occorre poi ricordare che il Governo ha adottato significative misure per l'innalzamento dell'importo delle pensioni più basse e che nel disegno di legge all'esame sono presenti misure riguardanti la totalizzazione dei periodi contributivi e il riscatto degli anni di studio universitari, che favoriscono le giovani generazioni. riguarda concerne il mercato del lavoro, l'eliminazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro intermittente costituisce la realizzazione di precisi impegni assunti con gli elettori, mentre la soluzione individuata con la revisione della disciplina sui contratti a termine ha il pregio di costituire un freno agli abusi, nel rispetto delle esigenze delle esigenze di flessibilità del lavoro, che non devono certo essere misconosciute. Sotto questo profilo, appare convincente ed equilibrata la soluzione individuata al fine di consentire la stipulazione di un ulteriore contratto a termine una volta superato il limite di trentasei mesi. Infatti, il rinvio alle parti sociali del compito di definire la durata del predetto ulteriore contratto e la previsione che esso venga stipulato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante di un'organizzazione sindacale adeguatamente rappresentativa, consentono una gestione della flessibilità in grado di scongiurare il rischio che essa degeneri nel precariato o nella violazione delle norme contrattuali in materia contributiva, come oggi avviene, penalizzando soprattutto le donne e i giovani. Vorrei inoltre ricordare le misure che riguardano la rimodulazione dei trattamenti di disoccupazione e la rilevanza delle norme di delega per il riordino degli ammortizzatori sociali, che puntano a porre fine ad ingiustificate tra i lavoratori legate esclusivamente alle dimensioni delle aziende presso le quali sono impiegati e ad estendere alcune tutele a lavoratori che finora ne sono stati privi. Vi sono, dunque, molte ragioni per sollecitare l'approvazione definitiva di un provvedimento come quello all'esame, che recepisce fondamentali richieste provenienti dal mondo del lavoro. Al tempo stesso, l'impegno del Governo sul versante sociale non può ovviamente esaurirsi con il varo delle norme che recepiscono il Protocollo del 23 luglio scorso.

Naturalmente, per tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, occorre procedere rapidamente al rinnovo dei contratti ed esercitare un controllo efficace sui prezzi e le tariffe. Gli altri temi di rilievo che dovremo affrontare nei prossimi mesi riguardano le iniziative di contrasto del precariato, affrontate anche in sede di ultima manovra finanziaria, e la prosecuzione dell'impegno già assunto con l'approvazione della legge n. 123 del 2007 sul fondamentale tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Rispetto a questo

sul lavoro. Ovviamente, l'impegno del Governo, per essere effettivamente ed efficacemente esercitato nei prossimi mesi, ha bisogno della fiducia della sua maggioranza. Ed è proprio per questa fondamentale fondamentale ragione che il disegno di legge va approvato dall'Aula nei prossimi giorni e con gli stessi contenuti concordati con le parti sociali.

Signor Presidente, colleghi, compagni della sinistra, io sono contrario, razionalmente e decisamente contrario, al Protocollo del 23 luglio Sono contrario e credo che i comunisti non dovrebbero mettere al primo posto la tenuta di questo Governo (sempre più subordinato agli USA, alla NATO, alla Confindustria e al Vaticano) sospingendo al secondo - o all'ultimo - posto le sofferenze, la miseria, persino la morte degli operai, dei lavoratori, delle donne, dei precari, dei giovani senza futuro. Sono contrario e credo che i comunisti dovrebbero votare no a questo accordo che umilia i lavoratori, toglie loro le speranze residue, approfondendo ancor più la distanza tra le forze di sinistra, il movimento sindacale e il movimento operaio complessivo. Sono contrario e credo che anche l'intera "Cosa rossa" dovrebbe votare no, e lo dovrebbe fare per nascere con un battesimo di lotta e non con la benedizione dei padroni. L'accordo del 23 luglio 2007, in verità, riassume l'intera legislazione del lavoro del Governo Berlusconi e, tradendo Seattle, tradendo Genova, l'intero movimento antiglobalizzazione, tradendo il milione di lavoratori del 20 ottobre, riassume la filosofia profonda della mondializzazione capitalistica: precarizzazione estrema, flessibilizzazione liberista, apologia di quel sistema capitalistico delle macchine che produce crisi continue di sovrapproduzione, trasformando gli esseri umani in pura merce di scambio, cancellando la garanzia suprema: Nella mia città, Ancona, gli operai comunisti del cantiere navale, negli anni '50, venivano facilmente licenziati; per sopravvivere facevano contrabbando di sigarette e con i soldi si ricompravano il posto di lavoro, pagando i dirigenti del cantiere. Oggi non riusciamo a sopportare l'idea che i lavoratori vengano di nuovo presi in giro, mortificati, che le loro minime garanzie sociali vengano sacrificate sull'altare confindustriale del Governo Prodi, sull'altare del ministro Padoa-Schioppa, un banchiere con il cuore di banchiere. Mi si dice, in modo sconsolato, perdente, che l'alternativa a questo Governo è la destra, è Berlusconi. Ma ci chiediamo (se lo chiedono ormai i lavoratori, l'intero popolo di sinistra): questo Governo è l'alternativa alledestre, a Berlusconi? Sappiamo, a partire dall'essenza delle cose, dall'essenza delle politiche, che non lo è, che il Governo Prodi non è l'alternativa a Berlusconi. Nasce da qui il pericolo grande della disillusione di massa, della stanchezza, della separazione dalla nostra gente, dal nostro blocco sociale, dai movimenti; anche da qui le basi materiali dell'antipolitica, dell'espansione molecolare dell'anticultura oscura della destra nel senso comune di massa; da qui la nostra possibile sconfitta strategica e la vittoria speculare delle destre. Noi non possiamo cadere nell'illusione di poter cambiare le cose attraverso queste sterili schermaglie da spadaccini istituzionali. Si è visto alla Camera come il tentativo di piccole modifiche sia stato frustrato dall'ala destra, sempre più in ascesa, dell'Unione, dagli uomini di Cordero di Montezemolo. Non vi sono alternative: le cose si cambiano a partire dal cambiamento dei rapporti di forza sociali, dal ritorno al conflitto. Il Protocollo del 23 luglio cala come un'ulteriore mazzata sul grande disagio sociale italiano, segnato già da sette milioni e mezzo di poveri e da otto milioni di persone che per cadere nella povertà hanno bisogno di poco: una rata del mutuo che non riescono a pagare, il rifiuto di un'altra cessione del quinto sullo stipendio, un figlio da mandare all'università. Credo di dire questo con cognizione di causa, non retoricamente, perché non è vero che il patto per l'Italia tra il Governo e i sindacati cancelli il cosiddetto scalone Maroni, ma anzi - con l'introduzione di nuovi scalini che prima non c'erano - allunga l'età pensionabile e peggiora le pensioni di anzianità soprattutto per le donne, costrette (da un dominio maschile che non cambia perché il mondo non cambia) non solo a lavorare in casa, ma a lavorare più a lungo in fabbrica e negli uffici. Vivo in una città dove le donne si alzano alle cinque di mattina, preparano il pranzo ai mariti, lo zainetto ai figli per mandarli a scuola; poi vanno in provincia (sino a sera, con un panino) a lavorare negli scantinati, a fare le camiciaie, per 600 euro al mese! Queste donne, queste lavoratrici, noi non le liberiamo, anzi allunghiamo loro l'età pensionabile. Queste donne, insieme ad un altro milione di persone, erano il 20 ottobre a Roma a una grande manifestazione di popolo che chiedeva di cambiare il Protocollo, che chiedeva di farla finita con le guerre e le spese militari: una manifestazione che tutti hanno celermente celermente e naturalmente dimenticato! Il Protocollo del 23 luglio non è solo controriforma pensionistica: in esso c'è la cancellazione di fatto del lavoro usurante, sino al punto che i poveri cristi che lavorano, si bruciano e muoiono negli inferni chimici e siderurgici non hanno più diritto a venir fuori qualche anno prima da quei *lager* della produttività e del profitto. C'è, scandalosamente, la ratifica della legge n. 30 del 2003, o legge Biagi, o chiamala come vuoi, tanto non cambia il senso: tu lavori quando vuole il padrone (tre mesi sì e sei mesi no; una settimana qua e l'altra là) senza più il minimo rispetto della tua vita, della tua sofferenza, del tuo futuro. La chiamano precarietà, ma è la consunzione di una vita, di milioni di vite, e i contratti a termine si allungano all'infinito. Nel Protocollo, dopo i tanti regali ai padroni, vi è anche la detassazione degli straordinari. Questa non si capisce proprio: attraverso gli straordinari degli operai, i padroni aumentano in modo esponenziale il profitto e su questo profitto extra (appunto, straordinario) non pagano tasse, mentre gli operai le pagano in modo esponenziale, poiché in un salario appena più alto aumentano i coefficienti e le trattenute sulla busta paga. Si tratta di salari di circa 1.000 euro, che sono tra i più bassi d'Europa e sui quali da oltre un quindicennio manca la scala mobile. Gli operai ammazzati dal profitto alla ThyssenKrupp erano alla quarta ora di straordinario, oltre le normali otto ore già passate in fonderia. Nessuno fa 13 ore di fila in fonderia se non per sopravvivere! A questi lavoratori viene trattenuta una quota fiscale sull'ora di straordinario, ma ai padroni no! Questi lavoratori, secondo il Protocollo, forse non fanno nemmeno più lavori usuranti. Questi lavoratori non possono andare in pensione qualche anno prima di morire. La loro morte ci fa soffrire, tutti, ma dobbiamo stare attenti alla retorica e alle parole scarlatte, che ho sentito anche in quest'Aula, tra la sinistra. Come per i soldati italiani in Afghanistan, si sta dalla loro parte in un solo modo: non piangendo dopo, dopo la loro morte, ma combattendo ora, per diminuire l'età pensionabile, ridurre l'orario di lavoro, alzare i salari, reintrodurre la scala mobile, allargare l'area dei lavori usuranti, abolire gli straordinari, perché i lavoratori debbono vivere degnamente, non giungere a 13 ore al giorno per sopravvivere. Sono contrario al Protocollo e credo che il Partito della Rifondazione Comunista dovrebbe votare no o, in subordine, votare la fiducia e ritirare poi la sua delegazione dal Governo. All'interno del mio partito e del mio Gruppo, con le mie forze, mi sono battuto per cogliere questo obiettivo. Lo stesso compagno e presidente Bertinotti ha dichiarato il fallimento di questo centro-sinistra. La possibilità di un mio voto diverso da quello del mio Gruppo non mi è concessa, pena l'espulsione. Ho parlato in questi giorni con gli operai di Mirafiori, con gli operai della Italcementi di Vibo Valentia, con i lavoratori della Telecom, e con tanti altri lavoratori e centinaia di compagni e compagne del mio partito. Personalmente non ho paura di nulla, nemmeno di un'eventuale espulsione, ma d'accordo con tutti loro devo continuare nel mio partito una battaglia politica ed evitare l'ulteriore diaspora di migliaia di iscritti e militanti. Credo che questo Protocollo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i miei colleghi (Roilo, Pegorer e Tiziano Treu nella sua relazione)

cominciare a valorizzare quello che di positivo contiene e le prospettive che apre, invece di confrontarci esclusivamente su ciò che divide. A differenza di altri colleghi, ritengo che il superamento dello scalone, la gradualità dell'innalzamento dell'età pensionabile, apra prospettive per un nuovo accordo tra le generazioni uscendo da una logica sbagliata e perdente riecheggiata anche in quest'Aula (per esempio, nell'intervento del senatore Baldassarri) che contrappone vecchi e giovani.

reale e sostenibile la svolta che esso segna rispetto alle politiche deregolatorie e neoliberiste che hanno caratterizzato il dibattito sul mercato del lavoro negli ultimi anni, per andare avanti e non restare fermi. Voglio farvi riflettere su un dato che, a mio parere, si pone alla base della sostenibilità o meno del nostro sistema pensionistico e incide sulla tenuta stessa del nostro sistema di *welfare*: è il dato che riguarda il tasso di occupazione.

Ciò che segna la differenza è la presenza o meno nel Paese di politiche di cura delle persone, di attenzione all'organizzazione del lavoro per garantire dignità e sicurezza.

capace di accompagnare i cambiamenti della vita lavorativa che sempre più frequentemente si porranno, qualunque sia il carattere e la natura del rapporto giuridico di lavoro.

Ecco, mi aspetto e mi auguro l'approvazione di una normativa europea e nazionale che tratti le persone come i fiumi, che imponga alle imprese l'obiettivo di far sì che ogni lavoratore che attraversa quell'impresa ne esca professionalmente impoverito ma professionalmente e culturalmente arricchito. Nella normativa, insomma, bisogna introdurre un nuovo diritto: il diritto-dovere di veder migliorate le proprie competenze professionali e culturali all'interno di ogni esperienza di lavoro. Per fare questo ci vuole davvero una nuova cultura del lavoro, decisiva anche sulle questioni della sicurezza di cui abbiamo parlato in questi giorni, perché alternativa a quella cultura dell'usa e getta, del profitto a tutti i costi che è alla base della insicurezza personale, morale e - ahimè! - anche fisica di gran parte del mondo del lavoro. Ed è questo - l'attenzione o meno ai processi di apprendimento ed alle persone - che decide la direzione verso cui marcia la stessa flessibilità, se è un modo necessario per gestire l'innovazione ed il cambiamento e innalzare la qualità del nostro sistema produttivo dei servizi o, invece, serve solo a realizzare, a costi minori, operazioni ripetitive e standardizzate all'interno di un sistema produttivo dei servizi che non sa compiere la svolta della qualità.

riprendendo magari Jacques Delors e la sua intuizione dell'Europa come continente della conoscenza, capace di tenere insieme competitività e coesione sociale. una verifica che, partendo da qui, renda possibile aprire un gioco non a somma zero, proponendosi di far crescere insieme cultura dell'impresa e del lavoro, ragioni della competitività e dei diritti: questa strategia ha negli investimenti in sapere e formazione il proprio punto fondamentale di connessione. Abbiamo due occasioni che spero siano al centro della stessa verifica di gennaio.

il disegno che ci siamo posti sulla riforma del *welfare* e dare un contributo a quel patto generazionale che è l'unico modo di risolvere i problemi strutturali di scarsa tenuta del nostro *welfare*. Un'altra occasione sarà la discussione cui il Governo si appresta a dar vita e che svolgeremo anche in Parlamento per rivedere, ridurre e semplificare gli incentivi per le imprese e diminuire contestualmente su di esse la pressione fiscale. È quella l'occasione per svolgere una discussione non rapsodica, ma per darci davvero una priorità che parta dalla difficoltà più grande che oggi

Per le imprese, perché la finanziarizzazione dell'economia rende sempre più necessari investimenti che si realizzano a breve e contrae i tempi di ammortamento degli investimenti; per i lavoratori, perché la compressione dei salari e il dramma delle tasche vuote dopo la terza settimana rendono difficile compiere investimenti per il futuro proprio e dei propri figli. per le imprese, per quel che riguarda la ricerca, abbiamo già uno strumento importante, il più potente che un Paese europeo abbia costruito: il 40 per cento di credito d'imposta per gli investimenti fatti insieme all'università e ai centri di ricerca, cui può aggiungersi un 15 per cento per gli investimenti in ricerca ed innovazione fatti in proprio. Credo che dovremmo compiere un ragionamento analogo anche in merito alla formazione, perché gli stessi investimenti in ricerca ed innovazione, se non accompagnati da una crescita professionale e culturale delle persone che lavorano, rischiano di non produrre quegli effetti d'innovazione tecnologica e culturale che auspichiamo. colleghi, il trasferimento tecnologico non consiste in macchine e forme, ma è fatto soprattutto da persone: la possibilità di una politica che trasferisca il valore della ricerca sulle imprese si basa sulla capacità e sulla possibilità di far crescere

signori del Governo, colleghi, vorrei partire innanzitutto da una considerazione preliminare, anche alla luce della relazione del presidente Treu che ha correttamente dato conto del dibattito svoltosi in Commissione e che ha cercato anche di fornire alcune risposte a due temi che, a mio avviso, però vanno approfonditi e chiariti. La prima questione: questo Protocollo è espressione di alcune parti sociali; questo è un Protocollo sottoscritto dal sindacato, dalla CGIL, dalla CISL, dalla UIL e da Confindustria; questo Protocollo lascia fuori pezzi importanti del sistema produttivo, determina una sorta di contrapposizione con il mondo del lavoro, in particolare del lavoro autonomo, lascia fuori tutti i soggetti, a prescindere dal riferimento d'area politica, dalla Confartigianato, alla Confesercenti, alla Confcommercio. Insomma, questo Protocollo non è esattamente espressione di una concertazione che tiene conto della nuova soggettualità all'interno della realtà italiana; è un Protocollo espressione di un segmento, importante, significativo, per carità, ma che pone uno straordinario problema che si chiama rappresentatività, soprattutto quando un protocollo così delineato e definito,

ma perché oggettivamente - come peraltro è stato riconosciuto con grande correttezza, da questo punto di vista, ed onestà intellettuale da tutti i colleghi della maggioranza, in particolare in Commissione lavoro la maggioranza non era in grado di affrontare neanche un voto su un emendamento eventualmente modificativo del Protocollo stesso. Ciò pone un'altra questione, ossia il problema corretto di un rapporto tra l'autonomia delle parti ma anche l'autonomia delle istituzioni, del Parlamento in particolare, nel compiere scelte che altrimenti corrono il rischio, al di là del merito della vicenda che stiamo discutendo, di eliminare un dato fondamentale, che è l'unico che dà senso alla politica; e la politica ha senso se si pone l'obiettivo di interpretare e di rappresentare il bene comune e l'interesse generale. Se non c'è questo, si pone attraverso meccanismi come quelli che stiamo affrontando e si dà paradossalmente un contributo ulteriore alla crisi della politica e delle istituzioni. Non abbiamo potuto discutere, non abbiamo potuto dibattere ed è una prima occasione persa perché credo che il confronto e il dibattito avrebbero consentito di approfondire un provvedimento significativo ed importante ed avrebbe consentito fin da prima un confronto più utile e qualificato. Lo dico perché noi abbiamo grande rispetto dei tanti lavoratori che nelle fabbriche hanno partecipato al *referendum* sul Protocollo. Avremmo però gradito se a quei lavoratori si fosse posta più di una domanda, non solo l'adesione al Protocollo, ma magari si fosse chiesto loro se ritenevano ritenevano che fosse più giusto il superamento dello scalone o se invece fosse più giusto mantenere sessant'anni ed in cambio, con quelle risorse, garantire più tutele, più protezione, più futuro per i propri figli. Non so come avrebbero risposto i lavoratori, ma non si possono costruire i meccanismi per adesione, per cui si fa il *referendum* per adesione e si fa persino il voto parlamentare per adesione, quindi il Parlamento è ridotto a sostanziale organismo di ratifica dell'accordo triangolare tra il sindacato, Montezemolo ed il Governo Prodi. Non credo si tratti né di buona concertazione, né di buona politica, né di buone relazioni industriali e, tanto meno, di buone relazioni istituzionali. Questo è quanto sul terreno dell'impostazione e del metodo,

È evidente che non si può fare un indistinto all'interno della vicenda del mondo del lavoro rispetto ai lavoratori ed all'età pensionabile. Tuttavia, proprio l'impostazione seguita dal Governo e dalle parti sociali che hanno sottoscritto il Protocollo ha determinato la prevalenza, sul terreno economico-finanziario, di una sola questione: quella del superamento dello scalone con gli scalini, diventata assorbente dal punto di vista finanziario tanto da determinare sia la difficoltà di individuazione e di copertura della platea dei lavori usuranti sia l'impossibilità sostanziale di cogliere l'occasione, non per mettere i giovani contro gli anziani,

Non ci sono oggi, se non aspettative rispetto a questa possibilità. Guardate: non mettiamo in dubbio che nel Protocollo e nel disegno di legge ci sono alcuni elementi positivi e se si votasse per parti separate noi stessi voteremmo, ad iniziare dal tema dell'indennità di disoccupazione, peraltro in continuità con l'impostazione del precedente Governo: viene aumentata un po' di più e spalmata un po' meglio, ma è in linea con il provvedimento già assunto dal Governo di centro-destra. Riteniamo che sia stato giusto affrontare il problema della totalizzazione, seppure in maniera ancora parziale, che però ha superato un limite che sicuramente impediva di utilizzare virtuosamente quel periodo lavorativo in termini contributivi e quindi previdenziali. Non siamo particolarmente convinti dell'impatto della misura sul riscatto della laurea, che per noi ha più valore mediatico - lo dico in senso positivo - che non in senso reale e sostanziale; non siamo convinti che sia giusta la strada dei fondi per l'accesso al credito o per quant'altro perché riteniamo che altre dovessero essere le misure Però, seguendo la logica per questa parte del provvedimento che pur dovrebbe dare contenuto a quel patto intergenerazionale, in realtà non possiamo tener conto di quanto è accaduto fino ad

Il lascito del Governo di centro-destra - vorrei dirlo alla senatrice Pellegatta con grande serenità - non è tanto lo scalone, ma il problema di un percorso di riforme incompiuto.

la riforma del mercato del lavoro, lo Statuto dei lavoratori, le nuove tutele ed i nuovi ammortizzatori, il tema della democrazia economica e della partecipazione. Il Governo di centro-destra ha determinato un pezzo di quell'*iter* di riforme e di cambiamento, che andava completato così come andava completato, sul terreno della riforma previdenziale, il tema del miglior utilizzo possibile, ai fini della costruzione della seconda gamba previdenziale, dell'utilizzo del TFR. del TFR. È lo stesso Governo che è intervenuto per utilizzare il salario differito dei lavoratori al fine di finanziare le opere pubbliche e le infrastrutture, non certo per consentire il migliore decollo possibile del TFR. Anzi, la fretta del recupero della risorsa finanziaria finalizzata a quel fondo ha determinato non già un meccanismo di partecipazione e di informazione ma piuttosto di dirigismo e di disinformazione, tant'è che non ci troviamo certamente di fronte al decollo di questo elemento fondamentale per la prospettiva, in particolare dei giovani, di una pensione più o meno adeguata. Il risultato di tutto ciò è che non diciamo con chiarezza alcune cose,

il tema della tutela dei precari, né la prospettiva della costruzione di un sistema di tutele. Infatti, in quel provvedimento l'indennità di disoccupazione continua a riguardare coloro i quali sono già garantiti, ma lascia fuori tutto il precariato vero, che non ha alcuna tutela. Da questo punto di vista vorrei dire al senatore Angius che ricordo il dibattito sulla finanziaria, l'ostinazione della componente socialista nel sottolineare questo dato, chiedendo, per esempio, che l'indennità, o un meccanismo analogo, fosse previsto per i Co.co.co. ed i Co.co.pro

le firme ad esso apposte, stanno nel segno del vecchio modello delle relazioni industriali, del vecchio modello delle tutele e delle garanzie, tant'è che non si affrontano le questioni vere che riguardano i veri precari precari e neanche il tema degli ammortizzatori. Diciamoci la verità, c'è una delega al Governo a realizzare entro dodici mesi la riforma degli ammortizzatori. Ma come e con quali risorse? A costo zero c'è scritto. È la stessa cosa scritta nella legge delega del Governo D'Alema, quando si fece una delega al Governo e anche allora, come oggi, con la pretesa di fare la riforma degli ammortizzatori

ed è per questo che la mancanza di confronto è ancor più significativa in termini negativi, perché bisogna confrontarsi non solo in termini di negatività reciproche ma anche di capacità di mettere in campo proposte diverse - ricordo a me stesso che il primo pezzo dell'indennità di disoccupazione è stato posto in essere in quel periodo. Ricordo a me stesso che risale a quel periodo il tema delle tutele per quei lavoratori delle imprese al di sotto dei 15 dipendenti, problema che è stato risolto, seppur in maniera derogatoria rispetto alla normativa vigente, attraverso un meccanismo virtuoso di coinvolgimento del territorio e della piccola azienda per determinare le condizioni utili a realizzare, per la prima volta, un'estensione di tutele che riguardasse non soltanto

Si trattava di continuare un percorso e di migliorarlo, non certo di stravolgere un'impostazione, che, ripeto, è così assorbente dal punto di vista della dimensione finanziaria che comporta anche un'altra questione, di cui hanno parlato e hanno scritto anche alcuni economisti di sinistra. Come si fa, dopo aver determinato un meccanismo in base al quale in dieci anni si spendono circa 7 miliardi di euro solo per il superamento dello scalone,

non fuori perché è evidente che alcune scelte di fondo vanno fatte. Il Governo ha fatto una scelta chiara e precisa, e quella scelta, Ranieri, non va in direzione del patto intergenerazionale,

che c'è chi disegna questo sistema come un sistema contro i giovani. Lo disegna in questo modo perché ai giovani stiamo sottraendo il futuro: il debito pubblico è infatti un furto di futuro.

come si fa a sostenere la tesi che questo Protocollo guarda al futuro se si aumenta la spesa previdenziale e non si utilizza, invece, l'occasione per rimodulare un'impostazione che vada in direzione delle tutele, delle garanzie e dell'inserimento nel mondo del lavoro? Rispetto alle cose che il senatore Ranieri ha detto noi non possiamo non essere d'accordo. È evidente che bisogna costruire e determinare un'impostazione che punti all'occupabilità per l'occupazione;

sull'inserimento nel mondo del lavoro rivedendo gli incentivi, determinando una serie di condizioni che soprattutto attraverso il coinvolgimento dell'università portino all'obiettivo fondamentale del trasferimento tecnologico che riguarda le persone.

e non affronta il tema di come determinare quella pluralità di soggetti del privato, del privato sociale e dell'università nell'incrocio tra offerta e domanda di lavoro perché anche c'è una differenza di ordine culturale. Noi guardiamo alla sussidiarietà orizzontale, voi avete legittimamente un'altra impostazione, sicché è difficile poi costruirle quelle politiche se si ha questo taglio e se si continua in tale direzione. È giusto affrontare il tema del diritto alla formazione come diritto individuale e della persona. Vi do atto che abbiamo già iniziato a farlo, seppur parzialmente, attraverso l'emendamento che io stesso ho presentato e che ha trovato la convergenza determinante determinante del centro-sinistra, ad iniziare dal presidente Treu, per inserire nella legislazione il diritto alla formazione - in quel caso per gli inoccupati come diritto alla persona finalizzato all'investimento in capitale umano, che è determinante nella conoscenza. Intendo dire perché gli interventi che ho ascoltato hanno rivoluzionato la scaletta che mi ero predisposto. È vero che dobbiamo ragionare sul tasso di occupazione,

Non si raggiungono quegli obiettivi senza un'accelerazione della crescita e dello sviluppo del Mezzogiorno. Il problema è che, anche attraverso la finanziaria, il Mezzogiorno non è centrale: ma non in quanto questione meridionale, come storicamente è stata affrontata e conosciuta, ma come questione nazionale riguardante il Sud come il Nord, in quanto riguardante il sistema Paese nella sua totalità e globalità.

Invece, è esattamente questo il modo per costruire l'alternativa da parte del centro-destra sul terreno dei contenuti e della rappresentanza sociale. Quindi, se dovessi concludere il mio intervento con una battuta

Se il Parlamento votasse su questo provvedimento, da destra a sinistra (a volte anche per qualche ragione condivisa), il provvedimento sarebbe bocciato. La verità è che con la fiducia a questo provvedimento si supporta e si tutela l'unico precario, cioè il Governo Prodi. Prodi e il suo Governo, invece, meriterebbero un licenziamento personale e collettivo perché non vi è fiducia parlamentare che tenga quando s'interrompe il rapporto di fiducia che

Signor Presidente, dall'inizio della legislatura, in ragione della rappresentanza voluta dagli elettori, il Senato della Repubblica opera in un contesto che sollecita e premia, soprattutto nella maggioranza, l'attitudine a differenziarsi, distinguersi e, talvolta, dissociarsi. Su una questione delicatissima per la maggioranza, quale quella in discussione oggi, vorrei tentare l'esercizio contrario. Vorrei cercare, nel Protocollo di luglio in materia di previdenza e di lavoro, una valutazione che possa risultare accettabile fra portatori di visioni differenti della politica sociale,

Data la consistenza delle parti sociali che hanno concorso alla formazione del Protocollo, e che poi si sono misurate sul risultato, e dati gli interessi primari che coinvolgono la generalità dei cittadini, si può ben dire che sulla approvazione della manovra finanziaria, di cui il Protocollo è parte essenziale, il riformismo è alla prova. Il Protocollo di luglio viene così ad essere il banco di prova dell'intera sessione di bilancio e di quella combinazione fra crescita ed equità sulla quale è fondato il riformismo della maggioranza precariamente uscita dalle elezioni del 2006. Ora, io penso (ma pensarlo è superfluo, perché si vede ad occhio nudo) che fra una concezione liberaldemocratica della politica sociale, quale la mia, ed una concezione radicalmente di sinistra l'arco sia molto largo e che arrivare che arrivare ad una linea condivisa richieda quasi sempre un compromesso. In ciò non trovo niente di male perché, come si legge nella teoria di Kelsen, il compromesso fa parte della natura stessa della democrazia. Nel caso del Protocollo di luglio, comprendente insieme alla previdenza norme importanti in materia di mercato del lavoro, di ammortizzatori sociali, di occupazione giovanile e femminile unitamente ad alcune misure per il recupero della competitività, il nodo del compromesso riguarda una questione cruciale da anni, e non solo in Italia, concernente il rapido prolungamento delle aspettative di vita l'opportunità di prolungare la vita attiva (anche in relazione alla diminuzione dei lavori più usuranti) e quindi un regime previdenziale sostenibile per le finanze pubbliche oltre che conforme a un principio di equità fra le generazioni. Il compromesso era (e parlo al passato perché il caso è risolto) il rispetto del contratto sociale stipulato dall'Unione con gli elettori, prevedente una correzione della chiusura a scatto delle pensioni di anzianità contenuta nella legge del 2004. Anche in ciò c'è un elemento di equità, nel senso che una drastica alterazione dell'età pensionabile al variare di un giorno introduce una sorta di lotteria sociale, senza altra motivazione che non sia quella casualmente anagrafica. A ciò si è provveduto con un innalzamento dell'età pensionabile più graduale e quindi più costoso, che peraltro sposta nel tempo, ma lascia immutata nella sostanza, la questione di fondo che è ineludibile: infatti, non si può ragionare di pensione di anzianità senza tenere conto di quanto sia diversa oggi, rispetto al passato anche recente, la condizione e l'idea stessa della persona anziana. L'imperativo per il bilancio nazionale è quello di adeguare il tasso di popolazione attiva tra i 55 i 65 anni agli*standard* medi europei e agli obiettivi dell'Agenda di Lisbona. Il Protocollo ha un costo quantificato, al comma 92, in oltre 10 miliardi di euro nel quinquennio dal 2008 al 2012. Questo costo si aggiunge agli oneri dei provvedimenti assunti con le due finanziarie del Governo Prodi e con gli altri ad esse collegati che, nell'insieme, rispondono ad una politica di redistribuzione dei redditi in favore dei ceti più deboli e degli individui più svantaggiati. Penso che si possa dire, anche in presenza di critiche autorevoli e non infondate, che l'intenzione redistributiva abbia prevalso nell'azione di Governo rispetto ad alternative anch'esse non meno apprezzabili, una maggiore riduzione del disavanzo pubblico e dello *stock* del debito, una riduzione significativa della pressione fiscale ed un maggior conferimento di risorse per rimediare al *deficit* infrastrutturale del Paese che sta diventando drammatico.

sufficiente per la sinistra antagonista. Ovviamente, sono in grado di offrire una risposta solo sul primo versante: la mia opinione è che in una democrazia liberale lo Stato non è soltanto il guardiano dei diritti privati, ma anche il soggetto che cerca di assicurare uno *standard* accettabile di vita a tutti i cittadini, perché un livello tollerabile nel tenore di vita finisce per essere la precondizione degli stessi diritti civili. Per applicarci alla presente condizione italiana, penso che l'azione redistributiva della mano pubblica trovi giustificazione oggi nella palese redistribuzione dei redditi verso l'alto verificatasi negli ultimi anni, gli anni in cui quel 2 per cento di abbienti che compongono la cittadinanza italiana ha notevolmente accresciuto la propria quota di ricchezza, mentre si è indebolita la capacità d'acquisto delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti e delle pensioni.

ma lo Stato può fare la sua parte, aprendo il sistema alla libera concorrenza; riducendo i ritardi nelle infrastrutture della modernità, quali quelle dell'energia, dell'ambiente e delle comunicazioni; liberalizzando i servizi a tariffa. In quelle direzioni, in un anno e mezzo, si è fatta meno strada di quella che era lecito aspettarsi. Dal momento che il nuovo anno si annuncia all'insegna della verifica, nel più vetusto lessico della cosiddetta prima Repubblica - che in realtà è la Repubblica di sempre - è sperabile che, per la competitività, la produttività e la modernità innovativa, si verifichi un processo più efficace. Stando alla questione di oggi, ossia l'esame della manovra finanziaria da concludere prima della fine dell'anno, non si può disconoscere che, nei vincoli imposti dal risanamento dei conti pubblici, l'azione redistributiva praticata dal Governo a favore dei ceti più deboli è stata il massimo possibile: e il massimo possibile dovrebbe essere considerato sufficiente anche dalla sinistra, che dei ceti deboli rivendica storicamente - come ha sostenuto anche recentemente il presidente della Camera

Senatore, mi sembra che il Governo sia presente in Aula e abbia preso buona nota delle sue parole.

però di poter intervenire, senza che ciò faccia ritenere esaustivo quello che potrò dire, per chiarire alcune questioni che sono state poste nel suo intervento.

Il decreto legislativo dovrà essere accompagnato da una relazione tecnica, fermo restando il principio, che viene ribadito, del rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

È doveroso che un così importante senatore si preoccupi di tali questioni. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, a mio parere, il fatto che tutti i dibattiti generali avvengano normalmente ad Aula quasi vuota che incita talmente all'intimità tra di noi che ci viene spontaneo darci del tu, come è successo al senatore Viespoli nei confronti di un altro collega - significa qualcosa sulla corporativizzazione del pensiero politico, ma di questo ma di questo forse si discuterà un'altra volta. Prendo volentieri spunto, parlando a nome del Gruppo di Rifondazione comunista e suppongo anche di altri colleghi della sinistra,

la più straordinaria forma di Stato che sia esistita sulla faccia della terra ed è una gloria del pensiero e dell'azione politica europea perché al di fuori dell'Europa questa forma di Stato non si è mai vista. È sicuramente anche uno degli sviluppi possibili della democrazia liberale e dello Stato liberale di diritto di cui giustamente il senatore Zanone si fa interprete. affermazioni fanno parte di quelle impropriamente definite né di destra né di sinistra e sono invece costituzionali e di cittadinanza. Questo è il fondamento generale. Non occorre mettersi d'accordo ed essere particolarmente benevoli e gentili gli uni verso le altre - cosa sempre gradita, ma non obbligatoria perché invece è obbligatorio che noi teniamo conto della Costituzione come terreno unico e del fatto che per la Costituzione noi siamo cittadini e cittadine. Ad esempio, una forma di Stato assistenziale, impropriamente definito *welfare*, ci riduce di nuovo nella condizione di sudditi perché chi deve chiedere qualcosa e non ha diritto di esigere il rispetto di un diritto soggettivo non è cittadino, mi spiace, ma un suddito che intraprende un rapporto di dipendenza, di gratitudine questa sì, obbligata - nei confronti di chi eroga qualche sovvenzione. Allora, se vogliamo tenere conto dello sviluppo del pensiero costituzionale, della definizione dello Stato (così come appare nella nostra Costituzione), si può dire che lo Stato di diritto che fonda la cittadinanza (ed è sicuramente un merito del pensiero e dell'azione liberale) può svilupparsi in vario modo, diventando, per esempio (questo è un rischio attuale), lo Stato delle società complesse, quale quello

veniamo catapultati al 1891‑1890. Dal 1890 al 1910 la grande democrazia liberale dell'Italietta (siamo abituati a chiamarla così, ma tanto Italietta forse non era) compì alcuni importanti passi in avanti sull'affermazione di una democrazia non soltanto formale e di cittadinanza puramente proclamata. Per esempio, predispose i testi unici,

Italietta). Istituì, inoltre, l'ente comunale di assistenza riferito a chiunque si trovasse sul territorio italiano, senza riferimento al domicilio di soccorso, in condizioni di bisogno. Dunque, un diritto soggettivo esigibile riferito a tutti gli appartenenti alla cittadinanza italiana.

studio. Gli sviluppi della medicina moderna consentono di guarire molte cose? Si rende necessario il diritto alla salute, al lavoro, alla casa eccetera. Sono tutti bisogni, non valori astrattamente definiti.

chi organizza e distribuisce la ricchezza sociale prodotta di carattere nobile, elevato, degno, non di dipendenza, di clientela - se vogliamo adoperare il termine politico che traduce la dipendenza sociale in relazione politica diseguale - da cittadino

Come dicevo, noi famosi briganti diciamo le cose che sto dicendo in questo momento allo scopo di far sì che la famosa verifica di gennaio - anche il senatore

della parte che qui rappresento, che nella verifica siano precisamente contenute le ridefinizioni di cosa si intende per Stato sociale, non dunque una riedizione del corporativismo antico nella forma moderna dello stesso problema. È noto che i sindacati, anche nel bel mezzo della più illustre civiltà liberale, furono ritenuti strumenti di pura eversione: erano vietati;

Prima di scriverla, diede luogo ad una grande consultazione di tutti i vescovi europei, i quali disposero tutti che bisognava condannare il sindacato e sostenere che era obbligatoria la corporazione. Quest'ultima non ignora il conflitto, ma ritiene che debba essere autoritariamente definito e risolto dall'intervento pubblico o da quello di chi, in qualche modo, dirige la corporazione con i due confliggenti allo stesso tavolo. La concertazione, forse, potrebbe essere la riedizione moderna di un pensiero corporativo, che peraltro - lo dico per quelli che eventualmente sono molto attenti alle definizioni autoritative della Chiesa - pensa di riferirsi a Leone XIII ed alla sua *Rerum* *Novarum*: in tale vanno bene le corporazioni ma il sindacato non è vietato. Allora, perché, a mio parere, dal punto di vista formale, definitorio e procedurale, questo decreto pende verso

propria funzione specifica, ossia varare le leggi: non è possibile che un Governo mandi in Parlamento un testo blindato. Lo stesso vale nei confronti della dialettica sociale:

a sé, ma che rappresenta in modo coerente un tassello della strategia con la quale il Governo Prodi, in questo anno e mezzo, sta governando con pazienza, determinazione ed ostinazione, al fine di portare fuori il Paese dal declino ed avviarlo sulla strada dello sviluppo, inserendo elementi importanti di equità. La seconda ragione è che la riforma Maroni aveva due elementi di debolezza e incoerenza. È giusto - anzi, è necessario - porsi il problema dell'elevamento dell'età pensionabile, ma il modo in cui tale innalzamento è stato adottato non non solo non era giusto, ma era anche repentino e brutale. Andavano introdotti - come fatto con il provvedimento - degli elementi di maggiore equilibrio e di maggiore gradualità, salvaguardando la specificità dei lavori usuranti. Il secondo lato debole della riforma Maroni era relativo ai problemi della flessibilità. ai problemi della flessibilità. Tali problemi, come si è dimostrato, si sono trasformati in precarietà ed era quindi necessario introdurre delle prime misure correttive, perché sappiamo benissimo che la precarietà non è solo un elemento di profonda ingiustizia per i giovani, ma è anche un elemento negativo per lo sviluppo, per la capacità, per la competitività del nostro sistema produttivo. Un lavoro precario non potrà mai consentire la realizzazione di lavori che abbiano elementi di professionalità. Quindi i correttivi che vengono introdotti creano delle condizioni per ridurre la precarietà e dare alla flessibilità il suo giusto significato e aprono la strada anche per operazioni importanti che devono riequilibrare nel settore degli ammortizzatori sociali.

dei provvedimenti e delle misure di carattere fiscale importanti (10.000 euro l'anno per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato al Sud; 5.000 euro l'anno per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato al Nord) perché riteniamo che l'azione debba essere congiunta e che il problema della precarietà debba trovare una soluzione.

con il blocco dei concorsi nella pubblica amministrazione, avevamo introdotto anche in quel settore, compromettendone l'efficienza, degli elementi inaccettabili di precarietà. Quindi, è un provvedimento che si muove sulla strada giusta ed è un movimento che completa e arricchisce la strategia del Governo, che oggi punta, con questo disegno di legge e con le altre misure che fanno parte del complesso della manovra di politica economica, anche a individuare soluzioni. Non sono parole al vento quando diciamo che bisogna intervenire sui salari e che bisogna aumentare il potere d'acquisto. di legge finanziaria all'articolo 1 abbiamo prenotato quelle che saranno le maggiori entrate che verranno dalla lotta all'evasione fiscale per destinarle ad un intervento rapido e forte che diminuisca il peso del fisco sulle retribuzioni dei lavoratori. Inoltre (lo rivendico perché anche nel centro-sinistra c'è sempre una tendenza quasi autolesionista di non valorizzare le cose che vengono fatte, c'è quasi un impaccio, una timidezza nel dire le cose che sono state fatte), per i pensionati abbiamo introdotto una misura particolarmente importante, per cui l'aumento che si è determinato per le fasce di alcuni pensionati contributivi sono, per la prima volta nella storia del nostro Paese, esenti da tasse, sono al netto e non incidono nella valutazione degli indicatori per avere i vantaggi degli interventi di carattere sociale. Quindi, abbiamo buone prospettive per dare una risposta al problema del potere d'acquisto e abbiamo buone prospettive perché sappiamo che dobbiamo combattere un fiscalismo che è eccessivo, dobbiamo realizzare sul serio un federalismo fiscale che non sia selvaggio, così com'è oggi nel nostro Paese, e sappiamo che dobbiamo affrontare con coraggio anche il problema di ridare efficienza alla pubblica amministrazione e che ci devono essere - come è previsto e come

che investe piuttosto che incoraggiare la finanziarizzazione della nostra economia. Questa strategia comporta la necessità di alcuni elementi di chiarezza, innanzitutto, nei confronti

per cui ritenere che le imprese siano tutte e solo rappresentate dalla Confindustria. Dobbiamo guardare con maggiore attenzione al mondo del lavoro autonomo, delle piccole e medie imprese, perché un problema di rappresentatività si pone anche per questo. Dobbiamo

inoltre, chiedere al mondo delle imprese di non fare il pianto del coccodrillo, ma di affrontare con decisione, assumendosi le responsabilità, i problemi della sicurezza. Abbiamo apprezzato le posizioni della Confindustria contro la criminalità e le posizioni prese, ad esempio, in Sicilia, ma chiediamo che sui problemi della sicurezza del lavoro vi sia un atteggiamento conseguente ed una presa di responsabilità

possono essere adottate solo sulla compressione del salario e su forme esasperate di precarietà perché queste sono ingiuste ed anche autolesioniste per il sistema delle imprese.

fatte da ultimo dal senatore Viespoli, quando ha assunto un atteggiamento dialogante ed ha espresso una serie di osservazioni che meritano una riflessione. Non condivido il ragionamento di fondo, alla base dell'intervento del senatore Viespoli, quando ripropone in maniera che ritengo stucchevole, la contrapposizione tra padri e figli,

non si chiudono con questi provvedimenti. Aprono un terreno di confronto sul quale è necessario che nel mondo della globalizzazione il futuro sia visto non come una condanna, ma come una opportunità

Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi già svolti dal presidente Treu e dai

invece, per quanto mi riguarda, questo accordo che è stato siglato con le parti sociali diventa ancor più importante e decisivo, proprio perché

L'elemento caratterizzante tale provvedimento è proprio quello di adottare, riprendendolo perché era caduto in disuso (forse perché non era moderno, come è stato detto), lo strumento della concertazione,

ad evitare pericolosi scontri; altrimenti, si parla di tentativi un po' spericolati, che rischiano anche di diventare disastrosi quando si mette mano a norme con le quali lo Stato cerca di eliminare disuguaglianze sociali a favore dei più deboli. Oggi non possiamo che sottolineare positivamente una svolta importante nel modo di governare, soprattutto quando si affrontano questioni forti e decisive per il Paese, vivendo momenti, appunto, di grande concertazione. Lo Stato sociale, le pensioni, il futuro dei giovani lavoratori sono certamente questioni difficili da governare, aspetti delicati e complessi del governo di un Paese. Non si può non dare atto è il frutto di un'intesa raggiunta grazie all'impegno che il Governo ha profuso in tale direzione e che ha messo insieme più di 40 associazioni, costituite da categorie sindacali e rappresentanze imprenditoriali.

interessi, un interesse comune. Come ho detto, questo accordo è stato ratificato dal voto di oltre 5 milioni di lavoratori e pensionati italiani, nei luoghi di lavoro e nelle fabbriche. Senza

Questo accordo raggiunto completa, con soluzioni coraggiose ed eque, la revisione del sistema pensionistico italiano. Non viene soltanto superato lo «scalone» introdotto della legge Maroni, ma altri risultati sono di straordinaria importanza, al punto da costituire un vero e proprio pacchetto di riforme: l'aumento delle pensioni più basse, legate ai contributi versati; la totalizzazione dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche; l'agevolazione del riscatto di laurea; l'aumento dell'indennità di disoccupazione; l'incentivo di secondo livello di contrattazione; e via dicendo. È un lungo elenco di questioni che consente di trovare

le condizioni per poter immaginare un percorso migliore successivamente. Dal punto di vista politico, l'intesa segna anche una svolta importante nel metodo, nei rapporti fra il Governo e il sindacato. Poi arriverò al ruolo del Parlamento dentro questa dinamica. Il Governo, mantenendo fede all'impegno assunto nel *memorandum*, ha scritto una pagina di concertazione complessa e difficile, ma importante; soprattutto ha stabilito, secondo me, un concetto di fondo:

con le parti sociali relativamente alle Ferrovie dello Stato e alla loro liberalizzazione sempre per favorire i soliti noti. Mi auguro che non sia così,

è stata l'idea tecnocratica della politica: il muro di posizioni retoriche, conservatrici e reazionarie, che miravano a non toccare niente o, al contrario, ad abolire tutto. Ha prevalso il senso di responsabilità nel Governo, così come nelle parti sociali. Il sistema delle quote, la vera novità, permette di recuperare maggiore flessibilità di uscita, ancorché ridotta nelle sue effettività potenzialità dalla soluzione tarpata che era stata imposta. Il principio è di quelli che consentiranno, nei prossimi anni, di salvaguardare l'impianto delle legge Dini che - ricordiamo - consentiva, ai fini della pensione contributiva, di scegliere a piacimento il momento del pensionamento dentro una «forchetta» compresa fra i 57 e i 65 anni tempo stesso l'intesa consente di superare l'*impasse* sulla revisione dei coefficienti di trasformazione. Concludo dicendo che questo cammino per arrivare all'intesa non è stato facile. Il sindacato, così come il Governo, ha dovuto guardarsi non soltanto dalle accuse di coloro che votano sempre contro distorcendo i fatti e negando le conseguenze positive delle misure introdotte a beneficio dei lavoratori e dei pensionati, ma anche dalle insidie di coloro che, ignorando i vincoli imposti dal quadro di finanza pubblica (e dagli impegni assunti dall'Italia in sede europea), hanno spesso minato le fondamenta della costruzione di un impianto socialmente e finanziariamente sostenibile. Molto resta da fare resta da fare per dotare il sistema di protezione sociale italiano di quegli strumenti che consentano, nel futuro sempre più immediato, di affrontare le grandi sfide derivanti dall'evoluzione del quadro demografico, dai cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dalle complessità di una società sempre più articolata e disomogenea nei percorsi di vita familiari e professionali. Ma la pagina scritta con questo accordo consente di guardare ai prossimi anni con maggiore fiducia; e con l'auspicio che sia possibile fare, e migliorare, i regolatori economici e sociali, senza contrapporre gli uni agli altri: i lavoratori attivi ai pensionati, i giovani agli anziani, gli uomini alle donne. PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Larizza. Ne ha facoltà.

per parlare di metodo, prima ancora che di contenuti, perché è uno degli argomenti trattati. Bisogna ricordare innanzitutto che se, il Governo e le parti sociali avessero potuto decidere senza il confronto fra di loro, probabilmente avrebbero scritto in modo diverso alcune parti dell'accordo. C'è stata, però, una scelta precisa del Governo, una scelta giusta di metodo e di sostanza politica: produrre queste riforme con il massimo consenso delle parti sociali. Per farlo, si è resa necessaria una mediazione che lo stesso Governo ha promosso e concluso, secondo me, con ragionevolezza, tanto da ricevere il consenso delle parti sociali, che pure rappresentano interessi diversi fra loro e, a volte, anche molto diversi. Nelle circostanze come questa, gli accordi sono possibili perché la mediazione sui contenuti è subordinata ad una regola imprescindibile: il Governo fissa l'agenda, conclude la mediazione e diventa garante dell'accordo. Il soggetto centrale è il Governo nella sua funzione istituzionale, che per definizione è unitaria e indivisibile. Un potere decisionale che si esercita in ragione di un preventivo rapporto fiduciario con la propria maggioranza. Non è un caso che la che la gestione della mediazione e delle sue conclusioni vengano da un impegno diretto del Presidente del Consiglio.

vi fosse la riserva di un secondo grado di giudizio "nella" e "della" maggioranza, nessun soggetto sociale accetterebbe di vincolarsi e sottoscrivere un impegno dagli esiti sconosciuti. Questo processo decisionale del Governo non può quindi che essere conclusivo, non solo perché è elemento di garanzia per le parti sociali, ma anche perché è la certificazione della credibilità delle scelte dello stesso Esecutivo. Alcune critiche sui contenuti, che oggi vengono avanzate al testo di questo accordo, possono trovare soluzione con norme integrative in una fase successiva per iniziativa diretta della politica. Dopo l'accordo, il sindacato confederale ha promosso una consultazione tra i lavoratori, i pensionati e i giovani, registrando una partecipazione e un grado di consenso molto elevati, superiori a quelli delle consultazioni precedenti. Sarebbe sbagliato non tenere in conto, nella massima considerazione, questa partecipazione e questo voto. Voglio ricordare che esso non riguardava i desideri del sindacato e del mondo del lavoro ma, esplicitamente e direttamente, i contenuti dell'accordo. un voto di consenso e sostegno pieno ai contenuti, cioè alla qualità della mediazione condotta dal Governo con il sindacato che ha sottoscritto

Rispettare e far rispettare i contenuti dell'accordo non è un punto d'onore del Governo, ma è una condizione politica decisiva, una necessaria garanzia che l'equilibrio raggiunto con le parti sociali non venga successivamente modificato a vantaggio di una parte o dell'altra dei contraenti. È chiaro che ciascun soggetto compie la verifica al proprio interno in corso d'opera, cioè durante le varie fasi del confronto e non alle sue conclusioni, affinché alla fine vi sia piena consapevolezza dei risultati. Il Governo ha promosso la riforma e ottenuto il consenso delle parti sociali perché la mediazione non era un preaccordo, ma un atto conclusivo condiviso dalle parti in causa. Solo la piena fiducia e la reciprocità dei vincoli con la propria maggioranza parlamentare poteva consentire al Governo di produrre questa riforma, che forse non renderà tutti felici, ma sicuramente fornisce risposte convincenti ad alcuni problemi urgenti da risolvere e inserisce validi elementi di innovazione nello stato giuridico e sociale dei giovani, ma non solo di questi. La fiscalità sulle retribuzioni, i trattamenti pensionistici, le norme sul mercato del lavoro e gli ammortizzatori sociali sono i piloni principali di questa riforma. La legge proposta corregge alcune norme precedenti e, soprattutto, introduce nuove e necessarie forme di protezione sociale, peraltro molto invocate e lungamente attese, in particolare dai giovani. Non è una svolta radicale, ma un fortissimo correttivo del percorso che stava corrompendo la necessaria flessibilità, degradandola nella precarietà sistemica. Se vogliamo offrire ai giovani la prospettiva di minori preoccupazioni per il loro futuro, sappiamo quale sia la tastiera su cui operare. ha creato con il concorso delle parti sociali le condizioni per cambiare il presente e ha indicato un percorso utile per il futuro, che potremmo integrare e arricchire se già oggi ci impegneremo a tradurre in legge e rendere operative le riforme già decise. A questo testo e a queste proposte di riforma, a mio avviso, bisogna rispondere - anche da parte di chi non è d'accordo

Se qualcuno, prima di parlarne, provasse a spiegare cos'è la spesa pubblica pensionistica, sarei un cittadino grato: infatti, a meno che con essa non si intenda il pagamento delle pensioni dei dipendenti pubblici, la spesa pubblica pensionistica è una truffa linguistica che viene usata per contestare provvedimenti di varia natura. Se i senatori consentono, io, citando una persona qui presente, farò un esempio per far capire meglio di cosa parli. Nel 1997 stavamo facendo gli ultimi aggiustamenti al nostro sistema pensionistico. In un incontro amichevole e riservato con l'allora ministro del lavoro Treu (ora senatore, qui presente), si discusse una specie di minaccia che ci precedeva ed accompagnava. I giornali italiani,

Quando si vuole contrastare una riforma o un titolo di una riforma, credo che bisogna usare argomenti convincenti e veritieri. Ecco, quello della spesa pubblica pensionistica non è un argomento convincente e veritiero, a meno che qualcuno non spieghi cosa sia

dove si è avuto modo anche di esaminare quest'atto complesso, ovviamente ridotto soltanto nella catalogazione del *welfare*, ma che in realtà riguarda temi più complessi come previdenza, lavoro, competitività. Un atto firmato, come hanno ricordato qui i colleghi, il 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali. Si tratta, a mio parere, anche di un provvedimento molto complesso, che intende mettere a regime il sistema pensionistico e riprende il tema delle pensioni, dandogli una certa stabilità. anche in campo azioni positive riguardo ai problemi dello sviluppo, dell'occupazione, con una serie di provvedimenti intesi a contrastare la precarietà. Un Protocollo siglato, rafforzato dal voto dei lavoratori che chiedevano meno precarietà e più certezza per il loro futuro, e soprattutto miravano ad assicurare un futuro certo ai loro figli. Ma quello di luglio a mio parere è stato un grande processo di partecipazione democratica, che ha validato la concertazione tra imprese, parti sociali e Governo. Non riesco a capire, a comprendere le polemiche di questi giorni. Possono essere di carattere politico, ma mi chiedo: possono mai sbagliarsi 5 milioni di lavoratori che decidono sul proprio futuro? Potevano mai essere d'accordo gli stessi lavoratori con il cosiddetto scalone? Non è certamente migliore la modulazione graduale nell'innalzamento dell'età pensionabile rispetto ad un meccanismo che porta bruscamente l'età pensionabile a 60 anni? Penso che su questo abbiano discusso i lavoratori italiani. Queste sono le domande che anche noi potevamo porci e sinceramente la risposta dei lavoratori è stata forte, convinta e rispettosa anche di una legge naturale: quella stessa legge secondo la quale i figli possano ricevere più di quello che hanno ricevuto i loro padri, e non il contrario degli ultimi anni. Questo tutela il patto tra generazioni e non certo il patto che era stato messo in discussione soprattutto negli ultimi dieci anni. Era ovvio che bisognasse riequilibrare il sistema.

sulla carta, come direbbe qualcuno, ma semplicemente onorato un nostro impegno elettorale come Unione: favorire le categorie più deboli, come i pensionati al minimo; l'*una tantum* per gli incapienti (i 150 euro al mese a persona che abbiamo garantito); gli incentivi alle imprese per le assunzioni; la stabilizzazione già dalla finanziaria dello scorso anno di oltre 350.000 precari del pubblico impiego; l'immissione in ruolo di 150.000 insegnanti; il *bonus* per il Sud. Abbiamo utilizzato maggiori entrate fiscali, non abbiamo distribuito condoni - non era questo che avevamo intenzione di fare e non lo abbiamo fatto - ma possibilità di sviluppo ed equità sociale. Anche noi del Partito Democratico-L'Ulivo ci siamo posti il problema di come affrontare il precariato, soprattutto al Sud, di come implementare politiche di pari opportunità per la crescita e la competitività del Paese. La precarietà - lo hanno detto qui in molti - non è solo una condizione sociale, è anche un disagio mentale e, senza dividerci su chi è più vicino ai precari (perché i precari non li scopriamo ora:

Certo, non sarà facile, perché la situazione ereditata è pesante, specie al Sud: una disoccupazione di otto punti superiore al Nord, un lavoro grigio sfruttato e sottopagato e un lavoro nero dove "salario", "tutela" e "sicurezza" sono termini oscuri. Nel provvedimento abbiamo inteso sanare soprattutto la piaga del lavoro intermittente, le forme contrattuali più precarizzanti - come lo *staff leasing* o il *job on call -* che esasperano il concetto del precariato e del lavoro flessibile. In questa direzione va la scelta della limitazione del lavoro a termine, che è stato uno dei nodi principali dello stesso provvedimento. Voglio ricordare anche qui le misure per i giovani: il microcredito, il sostegno all'attività, il fondo per il credito ai lavoratori autonomi, il riscatto dei corsi di laurea, il diritto alla formazione (che è stato qui più volte ricordato). ricordato). In questo provvedimento, però, vi sono soprattutto misure efficaci a sostegno del lavoro femminile. Già nella precedente finanziaria con il cuneo fiscale il Governo aveva cercato di incentivare le imprese che assumevano più donne; imposta, la scelta è stata più incisiva. Sono anni che le ragazze si laureano in maggior numero, sono più scolarizzate, hanno desiderio di affermarsi, di investire su sé stesse, di poter conciliare lavoro, carriera, famiglia, tempo libero e purtroppo restano indietro e al Sud non cercano più lavoro. Più incerto è il lavoro e più debole è il*welfare*; più le donne non lavorano, più le famiglie sono povere e più, purtroppo, si registra

come i servizi all'infanzia e il potenziamento di altri servizi come quelli di cura. È evidente che il diritto pieno al lavoro per le donne è possibile se si realizza un collegamento efficace tra mercato del lavoro e riforma del *welfare*. Lavoro e welfare:

per le riforme e le innovazioni di cui c'è bisogno. C'è stato subito un consenso nei confronti delle misure che rimodulano i trattamenti di disoccupazione e di estensione degli ammortizzatori sociali di tutela di particolari categorie che ne erano prive. Già nella finanziaria dello scorso anno - lo voglio ricordare - estendemmo la copertura dei diritti di malattia e di maternità ai lavoratori a progetto e agli apprendisti. Abbiamo aumentato la contribuzione previdenziale dal 18 al 23 per cento, determinando così un miglioramento della condizione previdenziale per i giovani lavoratori. Quello che stiamo votando, colleghi, è un provvedimento complesso, dove crescita economica ed equità sociale sono i criteri di azione. Essi, soprattutto, indicano un'inversione di marcia che ci risolleva dalla condizione di stagnazione economica a cui eravamo purtroppo giunti

erano in molti ad entrare nel mondo del lavoro e pochi ad uscirne perché l'invecchiamento era ancora agli inizi, ebbene lo Stato sociale e i modelli di *welfare* potevano permettersi di essere generosi.

la speranza di vita si è allungata, i cicli familiari sono completamente modificati, le famiglie si ricompongono, ma si sciolgono anche con più facilità, la vita si è allungata e pochi adulti sopportano il numero crescente di anziani. Tutto questo ha prodotto un mutamento della società e i sistemi di *welfare* devono adattarsi a questi cambiamenti.

Ciò significa che dovrà cominciare a lavorare intorno ai 25 anni e forse dovrà terminare intorno ai 70: una

e ormai la formula della coppia e della famiglia nella quale c'è un *provider* e c'è una persona che, viceversa, utilizza il reddito guadagnato per il consumo della famiglia non esiste più e perché una famiglia

forse meno stabile del passato, ma che dobbiamo in qualche modo stabilizzare o rendere meno precaria. Altrimenti rischiamo di avere una popolazione invecchiata che non avrà

propone una revisione dei coefficienti con il 1° gennaio 2010, ma mette in piedi una commissione che deve riconsiderare i criteri di

credo vada apprezzato l'indirizzo in senso universalistico degli ammortizzatori, superando la loro

diverso universalistico, per il sostegno del reddito e per il reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati. È stato fatto un tentativo nella legislatura precedente con il reddito minimo di inserimento. Quel tentativo è stato abbandonato. Penso sia sia tempo di riprendere questo argomento e mi auguro che nella delega si possa procedere in questa che è la direzione verso la quale tutti gli Stati moderni stanno andando. Importanti, credo, siano anche i provvedimenti che riguardano i giovani. Più volte ho insistito sugli aspetti drammatici della condizione giovanile di oggi, drammatici sia in senso oggettivo che soggettivo: in senso oggettivo, perché ormai rappresentano una risorsa sempre

rappresenti più e meglio di tutti lo stato confusionale in cui versa questa maggioranza. Così come più di tutti gli altri provvedimenti e meglio di tutti per il modo in cui perviene all'esame dell'Aula - rappresenta qual è stata la considerazione che questo Governo ha avuto e ha del Parlamento e delle sue prerogative. Vorrei ricordare, infatti, che questo provvedimento nasce fuori dal Parlamento, con l'attivazione dell'istituto della concertazione, fra l'altro, in questo caso poco rappresentativa sia per quanto attiene la rappresentanza sociale, sia per quanto attiene la rappresentanza datoriale. datoriale. Fuori dal Parlamento nasce un provvedimento a forte valenza sociale, economica, un provvedimento i cui temi portanti - il sottosegretario Montagnino lo sa bene per aver fatto parte nella scorsa legislatura della Commissione lavoro

Oggi questo Parlamento si vede costretto a ratificarne il contenuto dopo che è stata, di fatto, impedita qualunque attività emendativa sia al Senato, che alla Camera dove pure il provvedimento è passato in Commissione ma i cui risultati emendativi sono stati completamente disattesi al momento della presentazione da parte del Governo del maxiemendamento sul quale ha chiesto la fiducia. Cosa dire poi del Senato dove in Commissione non è stato possibile da parte nostra presentare, discutere e sottoporre al vaglio dell'approvazione un solo emendamento per l'ostruzionismo messo in campo dalla maggioranza, ostruzionismo fra l'altro - devo riconoscere - ammesso dagli stessi esponenti della maggioranza con un atto di onestà intellettuale? Tralasciando la considerazione

delle prerogative parlamentari meritino una riflessione. Penso che ne vada rivisto il percorso, perché non tutto può essere demandato a Governo e parti sociali, relegando al Parlamento un atto di tipo notarile. notarile. Vorrei poi sottolineare che, per quanto riguarda il contenuto, questo provvedimento rappresenta più di tutti il passato, il presente ed il futuro di questa coalizione di maggioranza,

madre di tutte le precarietà del mondo del lavoro, e lo scalone della legge Maroni, fonte di iniquità e ingiustizia fra i lavoratori. Rispetto ai tuoni di quella campagna elettorale,

- altro non è che una somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) dove vige ancora l'articolo 18 e non sono possibili licenziamenti collettivi. Si tratta, quindi, di un sistema di tutele ancora più consistente di quelle riguardanti il lavoro a tempo determinato nella grande industria. La legge Biagi l'aveva introdotto per dare risposta ad un sistema

imponendo vincoli di tipo sostanziale. Si vuole ridurre, con questa legge, la portata di tale istituto? Bene, il risultato sarà - com'è stato detto - aumentare il lavoro sommerso: aumentare il lavoro sommerso: questo il risultato dell'eliminazione dello *staff leasing* e della riduzione dell'istituto del lavoro a chiamata. Naturalmente, si registra ancora qualche passo indietro per quanto riguarda i servizi all'impiego, ove riaffiora il ritorno ad una visione centralista e statualista, quando si riafferma la centralità del servizio pubblico all'impiego. Ciò è in contraddizione con quanto avviene nel resto d'Europa, non solo nei Paesi scandinavi ma anche in Francia, Spagna e Germania, ove la conflittualità fra pubblico e privato viene superata e accantonata in una logica di sussidiarietà che vede il coinvolgimento, nella fornitura di servizi all'impiego, del pubblico e del privato, nonché degli attori sociali. la sostanziale tenuta della legge Biagi, la cui impostazione strutturale non è mai stata messa in discussione, a cominciare dal Governo, per passare attraverso la fase concertativa e finire alla Commissione lavoro della Camera, unico luogo dov'è stato possibile un minimo di discussione nel merito e di attività emendativa, azzerata - come dicevo prima nel momento della presentazione del maxiemendamento. La struttura della legge Biagi ha tenuto. Se la struttura della legge Biagi ha tenuto e non è mai stata messa in discussione, ci aspettavamo un minimo di autocritica

che essa ha assunto anche quando era opposizione in Parlamento nell'attività della scorsa legislatura, quando la legge Biagi in particolare è stata demonizzata al punto tale è stata demonizzata al punto tale da attribuire ad essa tutto il precariato nel mondo del lavoro. Bisognava fare autocritica, però ciò significava porsi in continuità con la legge Biagi; continuità con la legge Biagi significava e significa porre mano ad un nuovo sistema di tutele, ad un nuovo sistema di ammortizzatori sociali. Certo, vi è stato un aumento dell'indennità di disoccupazione, ma si tratta sempre e comunque di una logica risarcitoria, sulla quale strada noi ci eravamo comunque incamminati. Manca però un disegno strategico per un nuovo sistema di tutele, che in una società comunque flessibile protegga il lavoratore essenzialmente sul mercato del lavoro e non solo nel rapporto di lavoro. Vi è una delega al Governo, si dirà. Abbiamo poca fiducia in questa delega, ma non soltanto perché non abbiamo fiducia nella maggioranza, ma perché nel momento in cui si delega il disegno di nuovo sistema di tutela al Governo e si impone che l'emanazione delle deleghe legislative avvenga a costo zero, è evidente che riforme su aspetti di così grande rilevanza sociale non potranno mai essere effettuate a costo zero. Non altrettanto bene è andata in materia previdenziale; siamo in presenza di una vera controriforma. Infatti, mentre in tutta Europa l'età pensionabile aumenta con l'aumentare della vita media, in Italia si abbassa l'età per l'accesso alle pensioni di anzianità. Bisognava eliminare lo scalone, bisognava onorare una cambiale politica nei confronti dell'ala radicale di questa maggioranza, cambiare politiche i cui costi vengono scaricati sulle giovani generazioni, sui lavori atipici. L'eliminazione dello scalone con L'eliminazione dello scalone con gradualismo comporta qualcosa come 10 miliardi di euro, sostengono il Governo e la maggioranza. Noi diciamo che comporta qualcosa che si avvicina ai 14 miliardi di euro nei dieci anni.

Ci preoccupa il problema dei lavori usuranti - lo diciamo anche a seguito delle affermazioni del Sottosegretario - e non solo perché è stato eliminato il vincolo al numero dei trattamenti, perché riteniamo che una volta definite le tipologie di lavori usuranti, in presenza o in assenza di un limite imposto ai trattamenti, in presenza o l'assenza di un limite negli impegni economici, scatta un diritto soggettivo a cui l'INPS è tenuto a dare risposta.

pena il collasso dell'INPS, con conseguente penalizzazione della competitività del Paese. Per tutte queste motivazioni e per altre che non è stato possibile illustrare per brevità di tempo, annuncio

anch'io cercherò di toccare i punti più significativi del provvedimento nei pochi minuti a disposizione, perché ovviamente un'argomentazione complessiva porterebbe via molto più tempo di quanto ce ne sia a disposizione.

L'attuale maggioranza, durante la campagna elettorale e anche nell'anno precedente, aveva posto tale questione come uno dei cavalli di battaglia del proprio programma politico.

la politica ha memoria corta e conta quello che si è detto la sera prima a «Porta a Porta». Però, ricordo ai colleghi della sinistra intervenuti che effettivamente vi è stato un momento di concertazione

la disonestà intellettuale. Stiamo raccontando balle belle e buone. Quindi, anche su tale questione, se non uno spunto di riflessione un minimo di buon gusto da parte dei colleghi della sinistra a non dire cose che sono veramente altro rispetto alla realtà! L'altra questione fondamentale, come anche qui è stato ricordato, è che in sostanza si doveva annullare la legge n. 30 del 2003 perché, come si è detto, madre di tutte le negatività di questo Paese. A parte che ricordo ai colleghi che, quando è iniziato il Governo Berlusconi

di questa legge che ha agevolato l'ingresso al lavoro a moltissime persone, anche grazie - va assolutamente detto - alle questioni legate all'immigrazione, dove ovviamente un Governo, con all'interno la Lega, anche se *obtorto collo*, ha però regolarizzato le persone con un lavoro e non quelle sotto ai ponti, come aveva fatto la precedente regolazione della Turco e compagnia.

una Cosa rossa, senza dare troppo fastidio a Montezemolo che vi ha tirato la volata nel 2006, lo capisco perfettamente! Però, sottolineatelo un po' meno perché non fate una bella figura

A parte che nella maggior parte dei contratti dell'industria è già così. Sono nel mondo del lavoro e dell'industria e vi assicuro che oggi il 95 per cento dei contratti di lavoro, a parte qualche dettaglio, possano essere rinnovati solo due volte. Altrimenti, già lì si innesca un problema con l'Ispettorato del lavoro e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. È già così nella sostanzialità delle cose. Ammettendo pure che qualche contratto particolare non fosse sottoposto a tale questione, voi dite che lo si può rinnovare quanto si vuole - non so dove, però lo dite voi - per un massimo di tre anni. Dopo tre anni, il lavoratore, il datore del lavoro, l'ispettorato del lavoro e ovviamente (questo non può mancare, altrimenti cosa fa dalla mattina alla sera?) un rappresentante sindacale, si presenteranno in qualche posto e decideranno eventualmente di andare oltre i tre anni.

Però questo poi lo dirà la storia e lo vedremo dalle statistiche negli anni futuri. Circa la questione dello scalone noi non abbiamo mai detto, a partire dal ministro Maroni in avanti, che quella soluzione fosse perfetta.

approvò i conti pubblici italiani, che erano sotto stretta osservazione, dicendo che ci sarebbero stati comunque i tre anni successivi per valutare la questione e porre rimedio alla cosa, perlomeno negli aspetti meno presentabili. Voi, alla fine, cosa avete fatto? Il gioco delle tre tavolette.

sottolineato la questione in questi anni. E sottolineo questi anni, perché ricordo ai colleghi della sinistra che ormai mancano venti giorni alla fine dell'anno e il 1° gennaio 2008 è lì, tra venti giorni, ma era lì da tre anni e mezzo.

avete prima dimezzato e poi raddoppiato gli stipendi ai dipendenti pubblici; avete fatto tutte le riforme Bersani di cui nessuno ricorda assolutamente niente, salvo il fatto che adesso le Coop possono vendere le cibalgine; se se questo è il Governo della sinistra e dei politici che rappresentano gli operai stiamo freschi! Io sono figlio di operaio; quindi, capisco perfettamente il mondo che voi pensate di rappresentare, ma vi dico con grande tranquillità che voi con gli operai non c'entrate assolutamente nulla.

persone perché nessuno sa di queste quante, grazie per esempio alla riforma Maroni, avrebbero comunque continuato spontaneamente a lavorare, quante invece avrebbero voluto per forza andare in pensione o quanto altro si può dire su tale questione. Non era forse più semplice inventare qualcosa come incentivi, defiscalizzazioni, incentivi all'uscita, per cui ogni mese in più che si faceva dava origine a qualche premio in busta paga o altro? Di cose da inventare per risolvere nella sostanza il problema,

il concetto di fondo è che, senza fare una battaglia demagogica, se vi stava a cuore il destino di queste 190.000 persone le questioni da discutere e su cui ragionare sarebbero state molte altre. Non posso non ritornare su alcuni concetti che qualche collega della sinistra ha evidenziato.

Voi chiamate *welfare* un'assicurazione di Stato. Non è che i cittadini ricevano la manna come è accaduto nei 40 anni in mezzo al deserto, quando non lavoravano, andavano a letto la sera e, grazie ad un atto di fede, si alzavano al mattino e tiravano su la manna. Bisognava alzarsi presto sennò la manna si scioglieva come neve al sole. sole. Il *welfare* lo paghiamo in anticipo; la pensione non ce la regala nessuno: la paghiamo quando lavoriamo; la sanità non è gratis in Italia: si paga con le tasse; la scuola non è gratis in Italia: si paga con le tasse. L'unica differenza è che, essendo un *welfare* di Stato,

è esattamente come in Italia; la differenza è che il cittadino paga chi vuole e pretende ciò che vuole da chi preferisce. É una cosa diversa, dopodiché lasciatelo raccontare nei centri sociali che i "poveri negri" di Harlem se non hanno l'assicurazione vengono lasciati morire per strada perché chi va in America sa che non è così. Vorrei aggiungere: lasciate perdere questi discorsi perché purtroppo è così in Italia. Se arrivate al pronto soccorso un sabato sera e avete davanti 12 albanesi ubriachi che hanno fatto un incidente in macchina, voglio vedere chi manda avanti la settantenne con la peritonite che sta per morire. Ma questo è un altro concetto ancora. Per cui, smettiamola di raccontare balle.

tra quello che danno e quello che ricevono perdono 100 miliardi secchi di euro all'anno. Questo è l'unico Paese al mondo dove la gente paga obbligatoriamente per non avere indietro i servizi che nemmeno può scegliere. Quindi, anche su tali questioni la senatrice

la disoccupazione è diminuita e con gli incentivi fiscali modesti ma reali le imprese, in qualche modo, si sono rimesse in carreggiata e hanno riavviato un *trend* positivo.

perché era già evidente a tutti la pericolosa ritualità di questo dibattito che, in realtà, non è nemmeno più una discussione accademica ma, probabilmente, è un adempimento al quale siamo obbligati da alcuni barocchismi del nostro processo istituzionale.

ad affrontare quello che è uno dei temi epocali delle nostre società, cioè il rapporto tra vita di lavoro e vita di pensione e il costo rispetto alla collettività del prolungamento della vita media: tutti questi temi, connessi allo sviluppo e alla competitività, non riguardano solo l'Italia, ma sono affrontati oggi in tutto il mondo sviluppato, soprattutto sotto la pressione della globalizzazione e dello sviluppo di alcuni Paesi emergenti molto aggressivi su tutti i mercati. Questo tema dovrebbe

Non formulo alcun rimprovero nei confronti di chi non c'è, perché non occorre essere presenti dove è inutile esserci. Mi rendo conto che sto svolgendo un discorso parlamentare che ha lo stesso valore di un commento che avrei potuto esprimere durante un convegno o - dirò di più - di una conversazione che avrei potuto tenere a casa mia o in un bar con amici. I punti chiave del nostro dibattito non sono le cose che hanno detto, ad esempio, molti colleghi dell'opposizione, compreso il collega Galli - che ringrazio, perché ha usato molti degli argomenti che condivido - e i colleghi di Forza Italia: il il punto chiave è che stiamo dando prova, con una decisione preordinata che è quella di un voto di fiducia che non è stato chiesto ma si sa già ed è scritto dappertutto che si terrà in quest'Aula, che il Parlamento italiano non è un'istituzione

proclamano come virtuoso e democratico, perché non aggiungiamo la clausola che il Parlamento non se ne occupi? Per quale ragione occorre una legge per dare completamento a questo metodo? Non c'è ragione al mondo.

Non sono state delegate le parti sociali a decidere su quanto si dispone per legge; le parti sociali dovrebbero, nell'assetto costituzionale,

Esiste, in questo Paese, la cultura della concertazione che è antiistituzionale per sua natura, che esautora il Parlamento dai suoi ruoli, che attribuisce al Governo un ruolo di mediatore tra le parti sociali. Su tutto questo Confindustria e sindacati addirittura menano vanto di essere riusciti a raggiungere un accordo. Ma quanto più virtù repubblicana è stata dimostrata nella scorsa legislatura, quando il Governo si prese

di potersi rapportare rispetto ad un nuovo sistema previdenziale e per far fare le proprie scelte di vita in un tempo ragionevole, alla velocità che la globalizzazione e l'assetto economico mondiale richiedono nei cambiamenti della nostra società, anche per evitare che i nostri Paesi ricchi si avviino al declino, diventando Paesi impoveriti di fronte alla crescita dei Paesi emergenti, che sono gli unici, oggi, che producono ricchezza a tassi ragionevoli, oltre agli Stati Uniti. Quella seria assunzione di responsabilità repubblicana da parte di quel Governo e di quel Parlamento è stata accolta da tutti i protagonisti dell'accordo di oggi, in qualche misura, con l'idea e il retropensiero che tanto ci sarebbero state le elezioni, dunque si sarebbe potuto ributtare tutto all'aria e ridiscutere tutto da capo. È un Paese che può uscire dalle sue difficoltà e dalle sue crisi e diventare competitivo quello nel quale le riforme si accolgono con l'idea che possano essere smontate e buttate alle ortiche? No: è un Paese senza dignità. È un Paese senza dignità quello nel quale la maggioranza attuale conquista il successo risicato dei 24.000 voti, promettendo che abolirà alcune cose lo scalone, la legge Biagi e così via); in tal modo, raccatta un voto di tipo estremista, antisviluppo, di ribellismo sociale, di rivolta metropolitana e lo porta dentro il recinto istituzionale per prendere in giro solennemente quelle persone e dire poi loro che in realtà si farà un'altra cosa, fingendo di aver proceduto allo smantellamento delle riforme. Quando in

Ma voi, signor presidente Treu, avete uno straccio di dignità e di doti repubblicane per le quali non si sta almeno con chi ti dice che sei un assassinio, con lui non si partecipa alla stessa alleanza di Governo né si fanno ogni genere di forzature nell'ambito politico e parlamentare, dando un colpo al cerchio ed uno alla botte perché l'alleanza di Governo regga? Avete un minimo di sussulto di dignità per il quale vi rendete a catafascio questo Paese, con l'idea che, siccome siamo brutti e cattivi e non dobbiamo governare, voi vi potete alleare tra assassini e assassinati (perché questo è) e tra sfruttati e sfruttatori, e tra qualunque altra cosa vi possiate dire tra voi, pur di non essere

è il Governo che si assume la responsabilità ed è il Parlamento che decide, perché quello ha il mandato? Le parti sociali contribuiscono con idee, suggerimenti e proposte e discutono; alla fine, però, si decide qui dentro, perché qui risiede la sovranità popolare e non altrove. Se andate avanti così, porterete quella che definite l'antipolitica e che invece comincia ad essere la giusta indignazione di un popolo che vede una una politica imbelle ed inutile ed istituzioni di cui io mi vergogno di essere rappresentante, trovandomi qui a fare una discussione da bar (non per i toni, ma perché siamo ridotti ad essere come un bar). È giusto, quindi, che ci venga rimproverato di essere in qualche modo abusivi rispetto alla Costituzione, alla democrazia e alle legittime aspettative di un Paese che vuole cambiare, ma che voi state condannando al declino: declino: non volete neanche discutere delle leve che potremmo azionare per avviare il Paese in una direzione di sviluppo

con il maxiemendamento presentato dal Governo che include l'ormai famigerato articolo 1-*bis*. Abbiamo fondato motivo di credere - anche autorevoli membri del Governo si sono espressi in questo senso che tale articolo non stia in piedi perché il riferimento al Trattato di Amsterdam è errato e si riferisce ad un articolo che rende priva di senso tutta la formulazione dell'articolo 1-*bis*. La questione non ci preoccuperebbe particolarmente se non fosse che questo articolo è sostitutivo di una legge in vigore dal 1975: l'unica legge che punisce i reati di istigazione all'odio razziale, istigazione alla discriminazione razziale, discriminazione razziale, istigazione alla violenza per motivi razziali o religiosi e perpetrazione di atti di violenza per motivi razziali o religiosi.

che, tra l'altro, sono previsti da convenzioni e da trattati internazionali (non dal Trattato di Amsterdam, ma da convenzioni internazionali come, ad esempio, la Convenzione di New York contro ogni discriminazione del 7 marzo 1966). Il Governo ha fatto sapere, in modi del tutto impropri, cioè attraverso stringati e sibillini comunicati stampa rilasciati da singoli Ministri, che probabilmente il rimedio sarà trovato chiedendo alla Camera di approvare questa norma

quanto meno gentile da parte del Governo, oltre che rispettoso della Costituzione, farci sapere come formulerà questo comma nel cosiddetto decreto milleproroghe che entrerà immediatamente in vigore, anche rispetto ai tempi. se la nuova formulazione cancellerà alcuni di questi reati, tutti coloro che hanno commesso reati nel passato saranno automaticamente scagionati e non potranno più essere puniti; molte persone in carcere verranno liberate.

Avverto, inoltre, che alle ore 18 avrà luogo l'informativa del Ministro dei trasporti sulla protesta degli autotrasportatori e sui relativi effetti. I Gruppi potranno intervenire per non più di cinque minuti ciascuno,